nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la discussione sulla questione di fiducia. È iscritta a parlare la senatrice Brisca Menapace. Ne ha facoltà. Signor Presidente, componenti del Governo, colleghi, l'andamento di questo dibattito mette in luce alcune difficoltà che elencherò soltanto per titoli. Vi è innanzi tutto una difficoltà di relazione tra l'Aula e la comunicazione esterna: probabilmente anche da parte nostra sarebbe bene che assumessimo e mantenessimo un linguaggio più sobrio che non suggerisca alla stampa di dare conto dei lavori del Parlamento come se fosse un giallo, un *gossip* da settimanale femminile di quelli che si leggono dal parrucchiere. Anche da parte nostra mantenere un linguaggio più aderente alla caratteristica dei nostri lavori forse gioverebbe ed impedirebbe quelle

mi riferisco ad una protesta delle organizzazioni *gay* e lesbiche proprio perché, nel riferire della finanziaria, è stato messo in luce che, invece del testo concordato all'Osservatorio sulla violenza sessuale e di genere e contro gli orientamenti sessuali, quest'ultimo punto è caduto. Non credo che ciò sia avvenuto per malizia; del resto nell'espressione «violenza sessuale e di genere» può essere inclusa anche quella che riguarda gli orientamenti sessuali. Tuttavia il fatto che fosse stato concordato e sia saltato appare immediatamente come un qualcosa di sospetto. Credo proprio che dovremmo, per la prossima finanziaria, garantirci i tempi necessari anche per una stesura del testo che lo renda comprensibile e non equivoco. In ogni caso, protestiamo anche noi per questo questo non corretto riferimento ad una questione molto importante, almeno per conto nostro. Poiché si è anche le due Commissioni bilancio della Camera e del Senato non sono arrivate a concludere i loro lavori, credo bisognerà provvedere anche ad una modifica delle procedure per la composizione della finanziaria e sarebbe bene che questo progetto venisse affidato alla 5a Commissione del nostro ramo del Parlamento che ha così autorevolmente gestito e riferito sui lavori con piena soddisfazione generale.

per definire la Repubblica italiana ma, per l'appunto, il rispetto della Costituzione della Repubblica italiana. Il Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea è generalmente considerato, sia dagli estimatori che dagli avversari, un Gruppo molto corretto anche se ci vengono attribuiti poteri o capacità demiurgiche che non ci riconosciamo. Ad ogni modo, la correttezza ci è riconosciuta. Ciò dipende dal fatto che siamo quasi le vestali del programma;

dell'Unione ci teniamo molto che il metodo del consenso venga conservato anche perché esso giova alla composizione non imperialistica della volontà in un Governo di coalizione. A tal proposito potrei fare degli esempi. Quello Quello a me più familiare è relativo al casalingato. Probabilmente, un Governo di coalizione è come l'economia nel suo significato originario, che non ha bisogno di essere definita economia domestica della casa. Nel governo della casa bisogna mettere insieme età diverse, sessi diversi, diversi gusti alimentari, diverse capacità di resistere alle stagioni. Questo componimento

quando noi parlammo di discontinuità sulla politica internazionale fummo ripresi, ora l'onorevole Fassino afferma che la caratteristica di questo Governo dovrebbe essere proprio la discontinuità. Sono contenta di questa

Agganciata all'articolo 2 con legge ordinaria è la regolarizzazione richiesta delle unioni civili. Si tratta di cosa che non confligge. Queste due ragioni sono indipendenti, autonome;

Il cardinale non ha titolo per usare questi termini; deve pronunciarsi con termini rispettosi e, se ha delle difficoltà, può invocare un incontro specifico, ma non usare questi termini, poiché

*(FI)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, innanzitutto mi consenta un doveroso ringraziamento ai colleghi della Commissione bilancio che, nonostante la finanziaria sia costretta a passare con un voto di fiducia, si sono prodigati con grande impegno per portare taluni miglioramenti. Questa è una legge finanziaria pesante di quasi 40 miliardi di euro per obbedire ai *diktat* europei della Banca mondiale e del Fondo monetario. Ma, se contro le scelte del Governo si scatenano tutti, padroni ed operai, Sindaci di destra e di sinistra, qualcosa in questo Governo non funziona davvero. Ciò che colpisce di più in questa finanziaria è la sua straordinaria mutevolezza. Cambia ogni giorno. Ogni giorno compaiono e scompaiono tasse: tasse sui Suv, tasse sui motorini, tasse sulle automobili, tasse sull'eredità, tasse sugli immobili. Cambiano le aliquote dei prelievi fiscali per le varie categorie e corporazioni. Il *lobbing* di sinistra ha la meglio sulla politica. Difficile dire quale sarà la versione finale della finanziaria e solo all'ultimo voto si potrà dare un giudizio definitivo. Quel che è certo è che alla fine la vostra prima legge finanziaria sarà approvata con voto di fiducia. Solo dopo la finanziaria, quando entrerà nel vivo lo scontro a sinistra sulla formazione del Partito Democratico tra DS e Margherita, tomba di ogni residuo argine socialdemocratico, si capirà il futuro del Governo Prodi e delle residue speranze di un rinascimento italiano, come auspicato il giorno dopo le elezioni politiche da parte di molti esponenti dell'attuale Governo. Questa è la finanziaria peggiore della storia ed è originata da fondamentalismo ideologico. Infatti, è stata portata avanti con un dilettantismo quasi impensabile e viene approvata con un atto di arroganza e prepotenza che offende ancora una volta questa Aula del Parlamento. È una finanziaria una finanziaria iniqua, che toglie a chi ha meno, mentre ai ricchi non fa un baffo. Ai ceti medi fa pagare di più e rende quelli bassi ancor più poveri. Con questa manovra danno con una mano e tolgono con l'altra. L'aumento del bollo non riguarda solo le vetture di lusso, ma anche le auto medie. Sulla FIAT Punto, per esempio, citando dati del Ministero dell'economia, si pagheranno 180 euro in più. Certo, spero di essere smentito, visto che sui bolli c'è un tale caos che persino il vice ministro Visco ha detto che la colpa è del Parlamento. E qui non si capisce bene il perché. Altri fattori che peseranno sulle casse delle famiglie italiane sono l'aumento del riscaldamento, quello dell'ICI, gli effetti della revisione degli estimi catastali, i *ticket* sulle ricette. Insomma, in questa finanziaria non c'è equità, non c'è risanamento e non c'è sviluppo. Quella che il Governo si appresta ad approvare al Senato è una manovra finanziaria iniqua e sbagliata, che va riscritta di sana pianta. Ad affermarlo non sono io, cari colleghi: ad affermarlo senza mezzi termini è l'Adusbef, visto che saranno introdotte 56 nuove tasse che colpiranno tutti cittadini indistintamente. L'Adusbef ha tra l'altro stimato che un lavoratore con moglie e due figli a carico, con un reddito lordo di 37.000 euro, sarà tartassato da 226 euro di nuovi oneri. Riguardo poi ai persistenti rialzi dei costi di luce e gas, l'associazione non ha dubbi: occorre subito una liberalizzazione completa dei mercati locali delle energie, altrimenti il salasso ai cittadini è destinato a continuare. La manifestazione contro il Governo delle tasse e delle falsità, organizzata dalla Casa delle Libertà il 2 dicembre scorso, ha evidenziato il grave disagio che siete riusciti a creare in tutta Italia. È compito nostro dare voce e dignità a questa politica, allo scontento e al disagio che emerge dai ceti produttivi, che si sentono messi sotto tiro da una anacronistica, ma spietata vendetta di classe. Non c'è dunque tempo da perdere. In nome della rivoluzione liberale che saremo chiamati a portare a compimento dopo la parentesi del centro-sinistra che ci auguriamo breve, abbiamo il dovere di condurre un'opposizione ferma e responsabile sia nel Parlamento che nel Paese per bloccare la controriforma che il Governo Prodi sta cercando di mettere in atto, contro la quale tante categorie e tanti cittadini hanno dato vita ad una mobilitazione spontanea. Il Governo Prodi in sei mesi ha già battuto tutti i *record* negativi della storia della Repubblica. Ha trasformato l'Italia in una sorta di agenzia spionistica al servizio del fisco. È riuscito a far approvare dal Parlamento soltanto 13 leggi, ricorrendo per ben otto volte al voto di fiducia

Ha approvato alcune finte liberalizzazioni al solo scopo di far crescere i fatturati delle cooperative rosse, facendo venire allo scoperto un mostruoso conflitto di interessi sulle spalle del Paese. spalle del Paese. Ha portato ai minimi storici, e lo ha confermato l'OCSE martedì scorso, la credibilità dell'Italia all'estero subendo la bocciatura delle principali agenzie di *rating*. Ha dato un saggio della sua congenita incapacità con la peggior finanziaria degli ultimi cinquant'anni, una stangata iniqua e senza riforma. Ma soprattutto, record dei record, è crollato di 20 punti negli indici di gradimento. Un disastro senza precedenti di fronte al quale il signor Prodi chiede continuamente la fiducia del Parlamento perché sa di non avere più quella degli italiani. L'Unione tenterà di restare unita finché potrà, perché il potere è un collante eccezionale, ma nel momento in cui si accorgerà di non disporre più di una maggioranza politica

Per questo, a maggior ragione, occorre un impegno e uno sforzo eccezionali da parte di tutti noi affinché si realizzi una partecipazione nelle piazze, nei consigli comunali, provinciali e regionali. Dobbiamo dare un segnale di coesione e di forza all'Italia e un avviso di sfratto a questo Governo irresponsabile. Un Governo che tartassa così tanto come nemmeno il povero De Gasperi nel 1947, appena uscito il Paese da una guerra, riuscì a fare. Occorre dare un segnale forte, ma la forza ce la date voi, il territorio, la gente che produce, si alza la mattina, si rimbocca le maniche e comincia il suo quotidiano lavoro e sa cosa vuol dire risparmiare due lire per mandare avanti la famiglia. Ormai siamo arrivati al punto che alla terza settimana lo stipendio finisce. Siamo consapevoli che in Senato si combatterà una battaglia estenuante fino all'ultimo minuto, anche se credo che questo Governo e non cadrà certamente a breve. Ma la storia si ripete, cari colleghi. Teniamo duro che ce la faremo a mandare a casa questo Governo, costringendolo naturalmente ad implodere al suo interno.

dobbiamo tutti avere il senso del limite, dobbiamo riconoscere come non sia possibile consegnare ad una legge finanziaria il compito di cambiare il mondo, di mutare radicalmente condizioni sociali stratificate nel tempo, un compito in verità difficile da consegnare anche ad intere legislature ai soli Governi ed ai soli Governi nazionali. Ma da queste condizioni è necessario partire per segnare una visibile inversione di tendenza, per significare al Paese che è mutata la direzione di marcia. Da queste condizioni è necessario partire, non solamente perché questo è l'unico percorso capace di un corretto processo di emersione e di valutazione delle scelte, ma perché partire da ciò che è costituisce un dovere per chi aspira ad una politica non separata dalla materialità della vita quotidiana, dal destino concreto delle donne e degli uomini insieme ai quali vogliamo tentare l'azzardo di governare questo Paese. Parlare della situazione reale non è fuori tema, né fuori tempo, rispetto ai 1.400 commi della finanziaria, ai tanti colpi in battere ed in levare che vi si possono rinvenire e su cui sono puntualmente intervenuti i compagni del mio Gruppo. I dati di questa realtà non sono freddi e muti, sono al contrario capaci di irrompere nel dibattito che in questa Aula e fuori di qui abbiamo svolto, di fare giustizia delle tante grida che si sono levate anche oggi contro anche una sia pur minima manomissione del quadro esistente.

per cento sotto i 40.000 euro. Il 5,1 per cento dei contribuenti gode del 22,9 per cento del monte redditi. Vorrei chiedere ai colleghi dell'opposizione chi in questo elenco secondo loro appartenga al tanto nominato ceto medio.

con redditi intorno ai 70.000 euro, ma sono poco più dello 0,7 per cento di tutti i contribuenti. Ed il reddito non è tutto. La forbice si apre ancora di più se consideriamo la ricchezza che attraverso esso si genera trasformandosi in patrimonio e in rendita. La realtà è che viviamo in un Paese segnato da insopportabili squilibri. E' mutato nel tempo anche il modo di usufruire del reddito a disposizione. Qui, in questa città, ma in tutto il Paese, nonostante la flessione dei tassi di interesse, la conquista di un diritto essenziale come quello della casa è un miraggio. Negli ultimi quindici anni le annualità di salario medio necessarie all'acquisto di un appartamento sono più che triplicate. L'obiettivo irraggiungibile dell'acquisto di beni stabili si combina con la condizione di una crescente precarietà che spinge le ultime generazioni verso il prolungamento, questo sì a tempo indeterminato, signor Presidente, della dipendenza familiare e verso i beni futili. Assistiamo a nuovi fenomeni anche di difficile definizione, ad una sorta di inedita povertà consumistica. Lo stesso allungamento della vita media, che ha conosciuto negli ultimi cento anni un progresso per tutta la popolazione, rivela distorsioni profonde e, per la prima volta, una parte della popolazione, le donne a basso reddito, vedono diminuire la loro attesa di vita. Una destrutturazione che non solo attraversa e manomette gli equilibri economici, che non solo distorce la relazione tra la vita ed il lavoro, ma che aggredisce lo stesso rapporto tra presente e futuro, tra l'individuo e la società a cui appartiene. È questo ciò che ha sedimentato, e negli ultimi anni rovesciato, sulle nostre spiagge l'onda lunga della globalizzazione neoliberista. Difficile chiedere ad una finanziaria di mutare tutto ciò, impossibile non chiedere che cominci da qui. È la durezza di questo quadro che ci consegna una reale contraddizione: mentre ci induce a ritenere essenziali i passi compiuti, allo stesso tempo ci fa cogliere tutta la sua insufficienza. C'è davvero bisogno, signor Presidente, di un cambio di passo, ma non per mutare rotta, bensì per procedere con più coraggio, con più speditezza e senza ripensamenti notturni, sulla linea tracciata in quel patto con gli elettori che tutti insieme abbiamo sottoscritto.

- come viene ormai definito in questi momenti - il Governo dei fischi. Si fischia quando si va al Motor Show, si è fischiati quando si partecipa all'assemblea del CNA, si è fischiati per le strade anche della propria città.

Questo Presidente del Consiglio, che in questi momenti non è nemmeno apprezzato da quanti nella sua maggioranza lo sostengono, deve scendere in campo per difendere il super Ministro dell'economia e delle finanze; deve scendere in campo per sostenere che il suo Governo non ha bisogno di un suo secondo momento ma che tutto va bene in questo momento. momento. Penso solo alle università, penso ai rettori, signori del Governo, ai magnifici rettori che vi avvisano di non partecipare più a manifestazioni nelle università italiane, perché rischiate il fischio completo non più solo degli alunni, ma anche dei docenti, dei ricercatori, di quanti vivono ogni anno la ricerca e l'università.

ad una finanziaria che invece ha scontentato tutti, una finanziaria che non ha accontentato nessuna categoria sociale, nemmeno la più piccola in questo Paese. Una finanziaria di sacrifici, ma una finanziaria - come diceva ieri qualcuno dell'opposizione e qualche amico lo ricordava anche negli interventi di ieri sera - che impone addirittura

bianchi; tale operazione si poteva concludere con un accordo forte con le associazioni dei medici di base, prevedendo la possibilità di tenere aperti anche il sabato gli ambulatori medici affinché cittadini, che non avevano bisogno di cure ospedaliere, non si recassero in ospedale. Ma penso al recupero di queste somme, se è vero come è vero che, per esempio, una Regione come il Piemonte qualche anno fa introdusse il *ticket*

erano insufficienti a coprire la spesa che la Regione Piemonte aveva dovuto sostenere per tentare di recuperare il *ticket* sul pronto soccorso. È inoltre una situazione che torna ad essere ridicola, perché quando la finanziaria è arrivata in Parlamento si parlava del *ticket* sul

a carattere scientifico di avere responsabilità e di partecipare a convegni internazionali, perché gli viene vietato; mentre non viene vietato ai direttori scientifici delle strutture private e non viene vietato ad altri di partecipare a convegni. Allora, questa norma sulla finanziaria, la chiamerei con il suo nome, caro Presidente, con il nome del professor Cognetti, perché è la lotta della Ministra della salute al professor Cognetti.

per tentare di concludere il contratto del pubblico impiego per i precari. Vi faccio allora una domanda: questi soldi saranno sufficienti venti anni per coprire le spese del pubblico impiego o servirà un anno solo? Una volta sola si potrà attingere ai conti dormienti, una volta sola, e allora penso e ho paura, caro Presidente (finalmente è arrivato anche il Ministro dell'istruzione che di storie del precariato se ne intende), che non sarà possibile coprire per venti anni quanti devono lavorare in questo.

Il tentativo del Governo di non rispondere anche ad una serie di richieste unitarie della Commissione sanità (penso, ad esempio, ai talassemici e ad altri interventi che il Governo non ha garantito) ha posto in seria difficoltà

giorni fa in una seduta antimeridiana ho avuto modo di ascoltare il pianto del senatore Morando che, come Presidente della Commissione bilancio, si lamentava di non aver concluso l'esame in sede referente del disegno di legge finanziaria. Annunciava, nel suo pianto greco, implicazioni di carattere istituzionale allarmanti per i rischi sottesi all'approvazione della finanziaria da parte dell'Assemblea. Sono trascorsi appena tre giorni e come sempre il sistema ha trovato il modo per raggiungere gli obiettivi prefissati, in questo caso ponendo la fiducia. Quello che mi ha incuriosito, però, è che alla fine del suo intervento tutti i partiti, esclusa la Lega, come testimonia il resoconto stenografico, si sono accalorati nel battere le mani, pensando magari di poter risolvere con questa testimonianza la vera e grave malattia che inesorabilmente ha preso possesso delle istituzioni che rappresentiamo. Colleghi, sono entrato per la prima volta in Parlamento - non mantenendo però una continuità - nel lontano 1987: 20 anni fa. Il mondo esterno alle nostre istituzioni in questi 20 anni ha compiuto una rivoluzione tecnologica, e non solo, in tutti i settori:

Ascoltate gli improperi degli uomini della strada e capirete: queste scene fanno tanto pensare al Medioevo o alla monarchia. Continuo a chiedermi: ma non viviamo in una democrazia compiuta? Il principe, il monarca non ci Vorrei però tornare all'argomento del giorno, partendo dal pianto del senatore Morando: sappiamo che il pianto è la prima espressione che l'uomo compie quando viene al mondo. Mi auguro tanto che questo vagito sia il segnale per dare il via ad un progetto di riforme in senso federalista del Paese, a proposito del quale il Gruppo a cui appartengo è portatore di idee. Io in prima persona, nel 1987, alla Camera dei deputati proponevo questa linea federalista per il nostro Paese. Un concetto, però, che pochi conoscono e questa mia presunzione la leggo continuamente nei comportamenti e nei discorsi di tutti voi,

Mi sembrano cose di altri tempi. Parlando ancora della Commissione bilancio, il pianto era causato solo dalla mancanza di tempo per l'approfondimento dei vari articoli e nessuno ha pianto, escluso il sottoscritto,

vecchi, obsoleti per un Paese che si dichiara moderno. Questa è l'organizzazione di uno Stato centralista che rimarrà schiacciato dal peso della materia che continuamente attrae, arrivando poi ad implodere inesorabilmente.

perché obbligate a delle decisioni che vengono prese da un potere centralista. La finanziaria di un moderno Stato federale è limitata a pochi argomenti, pochi argomenti sono sinonimo di poco tempo, pur dando ampio spazio a confronti e a dibattiti. Mi sento, nella mia persona, anche uomo di grande responsabilità, mi rendo conto sempre di più che questo Paese, così com'è organizzato, è un gigante dai piedi d'argilla. Le manovre in atto sono sulla scacchiera politica del rifacimento di un'eventuale Democrazia Cristiana e questo mi mortifica, mi spaventa: il nostro Paese non ha bisogno di risuscitare non ha bisogno di risuscitare i partiti morti da tempo, che i morti seppelliscano i morti, un eventuale partito pronto al consociativismo è solo aberrante, anacronistico, oscurantista e servitore di *lobbies*, come è stato purtroppo per anni. Ho sempre servito e vissuto la politica come la massima espressione della carità, servono uomini di buona volontà; partendo da questo punto vorrei chiamare a raccolta uomini veri, che si sentono responsabili, direi doppiamente responsabili, come sono le regole del federalismo, cioè responsabili nei propri confronti e responsabili nei confronti della società, a cominciare un percorso di raffronto, di dialogo, per arrivare in tempi brevi a quelle soluzioni innovative per un Paese gravemente malato. Dal mio punto di vista, servono programmi e progetti intrisi di quei valori di cui la nostra società è testimone e depositaria, lontana dalle ideologie che tanto male hanno prodotto: solo così daremo un senso a questa legislatura, uscendo dagli schemi sterili per cui i senatori a vita permettono di poter arrivare a dei risultati. Il Paese ha bisogno di ben altre cose e, come ho detto prima, con programma e progetti chiari potremo arrivare a quei risultati che la nostra comunità, le nostre comunità e il Paese non possono più aspettare.

Signor Presidente, io voglio manifestare la mia soddisfazione, perché ho presentato un emendamento che riguarda le istituzioni che promuovono l'internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero e questo emendamento è stato accolto e recepito anche nel maxiemendamento. Ringrazio anche la sensibilità di molti senatori dell'opposizione, tra i quali lei stesso, Presidente, che ha posto la firma in questo emendamento. La La legge n. 549 del 1995 prevedeva cofinanziamenti alle istituzioni preposte all'internazionalizzazione delle piccole imprese, tra queste tra queste istituzioni vi sono le Camere di commercio italiane all'estero, che usufruiscono di circa un 40 per cento di questo capitolo. Con questo emendamento, con il quale ho richiesto maggiori fondi, che negli ultimi tre esercizi sono stati continuamente decurtati, quindi privando queste istituzioni della possibilità di svolgere la loro attività di internazionalizzazione delle piccole imprese, abbiamo recuperato risorse. La legge prevedeva che il cofinanziamento su progetti mirati fosse del 50 per cento, negli ultimi anni questi cofinanziamenti furono del 45, del 40 e ultimamente sono arrivati al 30 per cento. Era urgente recuperare questo aiuto che, ripeto, è solo un cofinanziamento su progetti mirati, il restante delle risorse vengono recuperate da questi enti localmente. Vorrei sottolineare, signor Presidente, che non è un emendamento che agevola gli italiani all'estero le Camere di commercio italiane all'estero -, ma prevalentemente le istituzioni italiane e le piccole imprese, che hanno tanta necessità di internazionalizzarsi, ed è un tema di continuo dibattito a livello economico, e includendo i consorzi che notoriamente sono un po' il fiore all'occhiello dell'esportazione italiana. Vorrei ricordare che siamo l'unico Paese al mondo

e sa quanto siano importanti e radicate sul luogo. Le Camere di commercio, in passato, hanno svolto addirittura funzioni diplomatiche.

In due mesi e mezzo abbiamo vissuto la costante trasformazione di questa legge sia nelle cifre (penso alle numerose tabelle presentate, rifatte e corrette) che nei contenuti, fra le proteste, i ricatti e gli ostruzionismi della maggioranza stessa verso il Governo, e, dall'altro, con le proteste certamente più nobili da parte di tutte le categorie del Paese. Un giornale ieri si divertiva persino a raffigurare il grafico delle cifre generali della manovra. A luglio, la finanziaria era anticipata dal Governo con un saldo di 35 miliardi euro; poi essa era approvata dal Consiglio dei ministri a 30 miliardi, divenuti dopo pochi giorni 33,4; il 9 ottobre erano 34,7, per effetto dei calcoli effettuati dagli uffici della Commissione bilancio della Camera; il 16 ottobre il saldo

Noi non abbiamo contestato solo il metodo confuso con il quale si giunge al voto di questa sera, ma anche e soprattutto i contenuti e prima ancora le cifre. Questa manovra non è né equa né solidale come il Governo si prefiggeva. Fra detrazioni e imposte indirette la fascia di reddito da lavoro dipendente che guadagna 1.300-1.350 euro netti al mese non solo non ci guadagna, ma perde qualche soldo e se a Torino i capi della triplice vengono fischiati significa che questa categoria di lavoratori non è sciocca e ha capito come funzionano le cose. I calcoli dell'ufficio studi della UIL - non del centro-destra - ci dicono che per chi si posiziona sotto i 1.000 euro netti al mese c'è finalmente un miglioramento di circa 6 euro netti al mese. Questa finanziaria poi non ha voluto minimamente tener conto delle maggiori entrate fiscali per il 2006. Le cifre iniziali del Governo sono inesatte. A fronte di 37 miliardi in più di entrate nei primi 11 mesi del 2006, il Governo ne ha riconosciuti solamente 26 e ne ha inseriti strutturalmente a bilancio - e dunque replicabili nel prossimo anno - solamente 5, considerando la rimanenza come occasionale. Se si considera che queste cifre non comprendono ancora l'autotassazione di fine anno, vi è la certezza che le entrate finali saranno ancora più alte. Queste maggiori entrate arrivano nelle casse dell'erario certamente non per la paura minacciata agli italiani da Visco nella caccia all'evasore, bensì per la lenta ma inesorabile ripresa che si avvertiva nel Paese insieme alla concreta crescita economica, contemporanee all'emersione dell'elusione fiscale, tutto ciò avvenuto grazie alle norme della precedente finanziaria. L'Esecutivo ha elaborato perciò una manovra vessatoria per i cittadini omettendo le cifre reali. Le ha omesse di conseguenza anche su quello che poi è il rapporto fra il *deficit* dello Stato e il PIL del Paese. Un *deficit* che, sempre grazie a quelle maggiori entrate, che potevano portare a una riduzione delle tasse, dovevano anche ridurre il *deficit* già al 3,2 per cento rispetto al 3,8 per cento previsto e contrattato da Tremonti con Bruxelles ad inizio anno. Ora, il Governo Prodi ha inciso in questa riduzione, secondo «Il Sole 24 ORE», solo per lo 0,03. Complimenti! Il resto è frutto della scorsa finanziaria. Invece, il Governo se n'è inventata un'altra: portare tale rapporto al 6

«Faremo ripartire il Paese», disse Prodi. Sì, ma con la retromarcia. L'effetto Prodi ha di fatto spaventato una ripresa economica già in atto. Noi a fronte di tutto ciò avevamo chiesto che con le maggiori entrate dell'erario si potessero apportare le seguenti modifiche al testo: sopprimere la revisione degli studi di settore, bloccare gli aumenti dei contributi per i lavoratori autonomi, bloccare gli aumenti sugli estimi catastali dei terreni, aumentare da 50 a 100 i dipendenti per il limite delle aziende escluse dalle norme sul TFR e, infine, stanziare almeno 500 milioni di euro in più per la sicurezza. Invece, tra emendamenti votati in Commissione e maxiemendamento, i benefici o meglio le toppe apportate al provvedimento sono stati ben pochi e peraltro accompagnati anche da peggioramenti. Tutto ciò è condito da una sequela di marchette, come correttamente le ha chiamate anche il collega Baldassarri, tanto per accontentare parenti e amici con la creazione di piccole e a volte inutili agenzie con finanziamenti a pioggia, dal Collegio d'Europa, al Museo della ceramica, al controllo delle nascite per cani e gatti o peggio col curioso cambio di nome ad enti come Sviluppo Italia solo per giustificare l'azzeramento dei consigli d'amministrazione. Credo che si debbano fare alcune considerazioni anche sui lavori della Commissione bilancio del Senato che, bene o male, per dieci giorni e dieci notti ha tentato di scalare la montagna di articoli ed emendamenti del Governo e della maggioranza. Vede, presidente Morando - purtroppo non è presente in Aula - lei ha ricevuto attestati di stima e riconosciuta correttezza da parte dell'intera Commissione. Il suo acceso intervento in Aula contro i metodi imposti dalla legge finanziaria, in un ingrato compito di portare il testo mozzato a causa dell'eccezionale numero di articoli voluti dal Governo, è stato applaudito anche dai banchi del centro-destra. Mi deve però consentire questa minima critica: mi sarei aspettato qualche parola in più nei confronti di un Governo che troppe volte l'ha messa in difficoltà senza dare risposte o dandole in ritardo alla Commissione.

Do atto della squisita cortesia al sottosegretario Sartor in Commissione, ma purtroppo è stata una scena spesso muta che ha comportato una fastidiosa laringite al presidente Morando, che alla fine ha dovuto parlare per tre.

Peccato che quella fosse una manovra da 26 miliardi, per oltre la metà composta di tagli veri. Erano altri tempi, che speriamo tornino presto, per la vostra salute, ma soprattutto per quella degli italiani. Questa finanziaria è stata accompagnata da tante bocciature: quelle istituzionali dell'OCSE e di tante agenzie internazionale di *rating* (per ultimo, la Standard & Poor's), oltre a quelle di molti economisti e quotidiani finanziari europei; ben più importanti sono state le bocciature del Paese. Caro presidente Prodi, i fischi e le contestazioni di un Paese che lei ha definito impazzito e che le fa pena non sono organizzati. Forse è lei che si è organizzato la *claque* qualche giorno fa, quando all'assemblea di un'organizzazione storicamente vicina alla sinistra è stato applaudito dai vertici di tale organizzazione. Provi a venire ad un'assemblea di artigiani veri, di commercianti o di imprenditori, ad esempio in quel Nord-Est dove l'intero blocco sociale del mondo del lavoro è totalmente contrario a questo provvedimento. nelle ultime ore sembra si sia aggiunto qualche ulteriore problema tra Fassino e Prodi su come interpretare la cosiddetta fase due dell'Unione. Noi suggeriamo una bella fase due: andate a casa prima di arrecare altri danni al Paese.

a chiedere sui fatti un'altra autorità indipendente, anche se ce ne sono parecchie, che certifichi al termine di ogni legislatura le condizioni del Paese.

nel modo più assoluto o a nascondere, attraverso un frasario con espressioni scarlatte, le condizioni nelle quali il Paese è stato precipitato dai Governi di centro-destra. Discutiamo se il peggioramento strutturale di saldi della finanza pubblica negli ultimi quattro anni abbia portato o meno il rapporto tra *deficit* e prodotto interno lordo a livelli inimmaginabili, che ci hanno fatto richiamare dall'Unione Europea; discutiamo se nel 2006, per la prima volta in dieci anni, non è aumentato il debito pubblico; discutiamo se il blocco pressoché completo delle risorse destinate agli investimenti pubblici non ha creato problemi e condizionato lo sviluppo economico del Paese.

ma non c'è dubbio che le condizioni generali del Paese sono peggiorate partendo da una regressiva politica di bilancio che ha colpito le categorie più deboli.

per così dire, cioè allo schieramento per il quale sono stato eletto in Senato). Certo, questo non significa - lo vorrei spiegare ai colleghi dell'opposizione presenti, ma anche a noi stessi

confederali. Vedete, si è parlato e si è scritto di fatti veri (che esistono e non sono stati inventati da qualche giornalista), della frammentazione della società;

Sono soldi dovuti! Ci dovremmo stupire del contrario e del fatto che - mi pare anche oggi o ieri - un grande istituto di ricerca abbia certificato che l'economia sommersa rappresenta un totale di 250 miliardi (se non ricordo male). Questi dovrebbero essere gli elementi di stupore, non il fatto che oggi vi siano è dovuto al Governo; è un fatto che ritengo rappresenti anche un elemento di eticità nel rapporto tra cittadini e Stato.

che si continua a parlare di sacrifici? Ho l'impressione - ecco, questo è un elemento di consenso sociale - che non si veda neanche la fine di questa galleria.

quella di cui (con espressione poco parlamentare: ma l'ha detto fuori di qui) il vice presidente del Consiglio Rutelli ha detto «chiamatela come vi pare, anche Topolino», il cambio di passo che ha chiesto anche il segretario dei facciamo in modo che questa fase 2 sia correlata alle critiche che abbiamo subito sulla finanziaria. Non vorrei che qualcuno

(mi avvio a concludere) ed è difficile spiegare la riforma se si aumenta l'età pensionabile e si diminuisce la pensione. Questa al mio paese si chiama controriforma pensionistica. Siamo stati votati per cambiare e questo dobbiamo fare, credo, in questi mesi.

dobbiamo anche sapere, e credo debba essere presente a tutti, che per le difficoltà della politica, del rapporto con la società, non ci sono scorciatoie. Possiamo avviare anche una riforma del sistema che impegna per sei mesi il Parlamento italiano a discutere di DPEF, bilancio e finanziaria, ma ci sono nodi politici che riguardano lo sviluppo e l'avanzamento della società, nella società, delle categorie più deboli e meno protette, nodi politici che dobbiamo porci come elementi per l'apertura di una seconda fase che porti a quel cambiamento il quale siamo stati chiamati a rappresentare molta parte del popolo italiano anche nel Senato. Presidente, onorevoli colleghi, in un certo senso l'intervento del presidente Caprili che mi ha preceduto è emblematico del teorema che sottostà a questa finanziaria e che, prima di entrare nel merito di alcuni argomenti, volevo commentare. Il teorema è quello di avere ereditato

Amato nel 1992. Ebbene, vorrei con pochissime battute commentare, presidente Caprili, e con altrettanta calma e serenità, quello che lei asserisce. Lei ricorderà come abbiamo ereditato il Paese noi e come invece lo lasciamo. Ereditammo il Paese con un buco finanziario riconosciuto per gran parte da voi stessi

Questi 19 miliardi di euro erano in parte dovuti ad errate previsioni sui ricavi delle tasse relative alla Borsa, perché fu un anno negativo per la Borsa dopo una serie

Una grande parte di questo buco era poi legata alla maggiore spesa sanitaria delle Regioni, scarsamente prevedibile *a priori*; un'altra parte (mi riferisco a circa 10.000 miliardi) era dovuta a manovre elettorali e a una finanziaria elettorale che aveva aumentato la spesa pubblica, quindi a spese sostanzialmente non coperte dai relativi ricavi. In sostanza, quindi, abbiamo ereditato un Paese con 19 miliardi di euro di buco. Come lo lasciamo complessivamente, presidente Caprili? È accertato ormai dal dibattito della finanziaria, e anche da quanto comunicato dal vice ministro Visco pochi giorni fa, che ci avviciniamo ad un *surplus* di ricavi, certamente dovuti allo Stato, che al 31 dicembre si avvicinerà ai 40 miliardi di euro.

che di questi 40 miliardi di euro 20 serviranno a coprire maggiori spese che si sono determinate all'interno di questo esercizio finanziario, noi vi lasceremmo comunque 20 miliardi di saldo attivo, cioè nei cassetti. Al contrario, voi ci avete lasciato 20 miliardi di euro di debiti.

di bugie - non saprei definirle diversamente - che si sono sentite in questi giorni in quest'Aula sullo stato dei conti pubblici ereditato

«Tra le opere sottoposte al CIPE, il 29,3% - sto riportando testualmente - risultano finanziate integralmente, il 51,1% sono dotate di finanziamento parziale, mentre il 19,16% sono approvate soltanto in linea tecnica». L'ammontare complessivo dei finanziamenti

il passato Governo nelle Ferrovie dello Stato ha speso 27 miliardi di euro, il precedente Governo - per fare un paragone di ordine di grandezza - 8 miliardi di euro. euro. Questo dà il segno dell'azione svolta dal Governo precedente. Bisognerebbe smetterla di dire falsità, autentiche falsità, sulla situazione ereditata dal precedente Governo. Ma questo il Paese lo sa benissimo e lo dimostra ogni giorno.

A mio avviso, manca ancora (ed è mancato soprattutto nella fase iniziale) un segnale forte di cambiamento di rotta a favore delle classi meno abbienti, di quei milioni di lavoratori e pensionati che non ce la fanno più ad arrivare a fine mese. In uno degli interventi di questa mattina

le pensioni dei lavoratori, in particolare le pensione più basse, hanno perso oltre il 34 per cento del potere d'acquisto, Paese si è verificato uno spostamento di ricchezza pari a oltre 50-60 milioni (oltre 100 miliardi di vecchie lire) dalle classi più basse alle classi più ricche, da quelle classi cioè che in questi anni hanno visto arretrare drasticamente le loro condizioni economiche e sociali. Inoltre, voglio esprimere grande preoccupazione su alcune intenzioni già palesate, alcuni appuntamenti già previsti in primavera che, se non correttamente gestiti, rischiano di dare un ulteriore taglio, peggioramento delle condizioni delle classi più deboli. Mi riferisco in particolare al tavolo già previsto sulle pensioni, alle questioni relative alla revisione della normativa sul mercato del lavoro ed alla rivisitazione degli accordi sulla politica contrattuale famosi accordi 1992-1993) relativi alla concertazione rispetto ai quali già da mesi Confindustria rivendica una ulteriore stretta sui salari, sui diritti dei lavoratori ed ulteriori aumenti di flessibilità della prestazione, attraverso quello che eufemisticamente il presidente di Confindustria chiama un nuovo patto d produttività e di sviluppo. Voglio dirlo con chiarezza: il mio partito ed io personalmente, ma anche credo a nome del Gruppo, ci batteremo con forza e non accetteremo che si vada nuovamente ad un taglio dei rendimenti delle pensioni, in particolare per le pensioni in essere ed in particolare che si metta in discussione il diritto per i lavoratori - mi riferisco in modo particolare ai lavoratori della produzione, ma anche a quelli dei servizi - alla messa in discussione del diritto di andare in pensione dopo una vita di lavoro con 35 anni di contributi e 57 di età. L'ho già detto altre volte. Voglio ripeterlo: i conti, per quanto riguarda il Fondo relativo ai lavoratori dipendenti sono in pareggio. Altri conti gravano sui costi generali del nostro sistema pensionistico. Non si può continuare a chiedere che i lavoratori dipendenti continuino a pagare per altri. Ciò premesso, voglio esprimere un forte apprezzamento per le modifiche contenute nel maxiemendamento sui temi della precarietà e del lavoro, così come i segnali di miglioramento che ci sono stati sui temi dell'ambiente e di uno sviluppo ecocompatibile, anche se devo rammaricarmi,

che, così come formulato, stravolge profondamente un principio sul quale si era convenuto relativamente al CIP 6. Chiediamo quindi al Governo di intervenire essendo conseguenti agli accordi assunti. In particolare, voglio esprimere un apprezzamento sui risultati conseguiti, sul tema della lotta alla precarietà, tra cui voglio citare il Fondo per la lotta al precariato nella pubblica amministrazione che, a mio avviso, non risolve tutti i problemi, ma potrà dare un forte contributo e risultati positivi. Ma nondimeno va apprezzata l'estensione dei diritti e delle indennità di malattia, in particolare per i Co.co.pro. e l'impegno del Governo per l'estensione del diritto alla maternità a rischio per queste lavoratrici che oggi ne sono escluse, cosi come l'affermazione di alcuni importanti princìpi in difesa del salario, quale quelli contenuti nel comma 774 che stabilisce due princìpi: l'aumento dei contributi, previsto in finanziaria, dal 19 per cento al 23 per cento non possono essere a totale carico dei lavoratori, così come è intervenuto la volta scorsa.

di reddito all'anno sono passati a 10.500 euro. Inoltre, tale comma stabilisce un principio per me importantissimo, che modifica decreto legislativo n. 276 del 2003, cioè che il trattamento economico di questi lavoratori deve far riferimento, rispetto alla professionalità che erogano, a quanto previsto nei contratti di lavoro.

perché non hanno una certezza e una sicurezza di lavoro e non hanno il reddito sufficiente per poter programmare una loro vita e costruirsi una famiglia. Infine, ed è l'ultimo punto che mi preme sottolineare con molta soddisfazione: credo che le misure che abbiamo introdotto in tema di potenziamento dei servizi per la tutela della sicurezza e altre norme

all'evasione, al lavoro irregolare ed alla non applicazione delle norme antinfortunistiche del

che favorisce le aziende che adottano i piani per la sicurezza, che applicano *in toto* le norme del decreto legislativo n. 626 e che non abbiano avuto infortuni, è un grande principio che può permettere di di avviare un percorso virtuoso per cui in fabbrica e nei posti di lavoro morire o avere infortuni non sia più una triste fatalità. Infine, ha un valore assolutamente emblematico, ma non per questo non importante, l'istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di gravi incidenti, soprattutto quelli mortali sul lavoro.

questa piaga che abbiamo nel Paese - deteniamo il primato in Europa sugli infortuni e sulle morti sul lavoro, cosiddette eufemisticamente morti bianche giorno muoiono mediamente tre lavoratori. È un percorso che in questa finanziaria stiamo avviando. Si tratta a mio parere di un primo pacchetto concreto di strumenti che da domani aiuteranno meglio il Paese e le istituzioni nella lotta per la difesa del diritto alla salute e alla vita nei luoghi di lavoro. Abbiamo risposto anche positivamente all'appello del Capo dello Stato, che più volte ci ha in questo senso invitati; ha invitato le istituzioni e il Parlamento a fare qualcosa perché questo fenomeno si contemperi e cessi e soprattutto per creare un clima nel Paese - perché di un clima nel Paese bisogna parlare - in cui il senso comune passi dal considerare oggi

alcune prime risposte significative in tale direzione. Per queste motivazioni, fermo restando il giudizio più complessivo, e fermi restando la volontà e il principio di continuare a batterci perché nell'azione del Governo si vada verso il pieno rispetto e l'attuazione degli impegni che abbiamo formulato nel programma comune, ripeto, anche sulla base di queste considerazioni, il mio voto sarà un voto non di disciplina ma un voto convinto.

Signor Presidente, signor Ministro, Sottosegretari, onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito della manovra, vorrei parlare del metodo utilizzato per elaborare la legge finanziaria. Nell'opinione pubblica, questa legge di bilancio è stata definita una finanziaria dalle porte girevoli; il Paese ha assistito una grande gestione molto confusa. La manovra cambiava di giorno in giorno creando insicurezza e malcontento nel Paese. Non hanno protestato solo gli elettori di centro-destra che sono scesi in piazza il 2 dicembre, ma anche gli operai della FIAT, il mondo universitario, i liberi professionisti, la base dei sindacalisti. La manovra - bisogna dirlo con franchezza - ha scontentato un po' tutta la popolazione, perché, con l'intento di accontentare tutte le categorie, si è raggiunto l'esatto opposto. Lo dimostra, purtroppo, la caduta del consenso di questo Esecutivo, una caduta che va messa in relazione ad una finanziaria troppo pesante e troppo fondata sulle entrate. Lo scontento che attraversa vari strati del Paese ci deve fare riflettere e non va sottovalutato. Ho già detto che, a mio avviso, una delle cause è stata la gestione confusa di questa manovra. Un altro aspetto che ha sicuramente deluso soprattutto l'elettorato di centro-sinistra è stato il mancato coraggio, ovvero l'incapacità di questo Governo di procedere con passo sicuro sulla via delle riforme economiche che il Paese produttivo si attende. Riguardo alle scelte coraggiose, accolgo con favore, ad esempio, la riduzione della spesa della politica, ma allo stesso tempo occorreva penalizzare nel pubblico impiego l'inefficienza e premiare la produttività. Sostengo la lotta all'evasione fiscale ma, al tempo stesso, critico un programma antievasione che prevede soprattutto ulteriori oneri burocratici che penalizzano in prima linea le piccole imprese. Esse costituiscono la larga maggioranza delle imprese italiane e il loro rilancio costituisce la condizione essenziale per la crescita economica di questo Paese. Il Governo ha giustificato l'entità di questa manovra spiegando che c'era da tappare l'ingente buco nei conti pubblici lasciato dal precedente Governo. È vero, la finanza pubblica andava assolutamente rimessa in sesto e gli sforzi dell'Esecutivo per il risanamento sono da apprezzare, perché non c'è dubbio: senza risanamento non c'è crescita. L'Italia non può più permettersi declassamenti da parte di agenzie internazionali. Occorre riconquistare la credibilità. Sostengo pertanto pienamente l'obiettivo di risanare i conti pubblici. Ma mi sarei augurato - e questi moniti vengono anche dalla Commissione europea - una maggiore riduzione della spesa pubblica. Entrando nel merito della manovra finanziaria sulla quale siamo chiamati a votare, intendo sottolineare che il testo originario aveva sicuramente bisogno di modifiche migliorative. Grazie all'impegno politico profuso nella cabina di regia e al lavoro in Commissione - che non è stato invano, visto che molte modifiche apportate in sede di Commissione sono state recepite nel maxiemendamento abbiamo raggiunto sostanziali miglioramenti al testo originario. Alludo, ad esempio, alle misure più *soft* per gli studi di settore, al passaggio delle imprese e franchigie disposte per i trasferimenti per successione e donazione tra coniugi e parenti in linea diretta, fratelli e soggetti portatori di *handicap*. Alludo anche ai ritocchi alla disciplina delle società non operative, all'esenzione fiscale dei contributi ENPALS per gli artisti dilettanti, all'estensione alle emittenti radiotelevisive locali di minoranze linguistiche dei contributi che spettano alle testate locali, e così via. Sono state introdotte delle novità delle novità interessanti anche per il settore ambientale. A tal riguardo, mi preme dirlo, non capisco come mai il Governo non abbia mostrato la necessaria sensibilità per il Parco nazionale dello Stelvio, il più grande dei parchi storici italiani e tuttora il più esteso dell'arco alpino. Come noto, infatti, il Parco dello Stelvio è retto, in forma consortile, tra lo Stato, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia. Vista questa situazione speciale di gestione, avevamo richiesto che i fondi regionali e provinciali di tale Parco non fossero soggetti alle limitazioni previste per le spese statali. Il nostro intento era garantire i rapporti di lavoro dei dipendenti, le misure già introdotte, nonché il rapporto complessivo sull'attività svolta. Mi rincresce molto che questa richiesta, tesa soprattutto ad avvicinare il Parco nazionale agli abitanti, non sia stata recepita. Colgo l'occasione per annunciare in questa sede che il Gruppo Per le Autonomie presenterà a breve un disegno di legge per risolvere definitivamente questo problema. A tal riguardo, chiediamo fin da ora l'appoggio del Governo per risolvere la questione. Concludo annunciando comunque, per i miglioramenti raggiunti, il mio voto favorevole a questa finanziaria. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, vorrei utilizzare il mio tempo a partire da una riflessione di ordine generale, da una sensazione. Ci troviamo di fronte ad una manovra enorme, di grande significato e di grande impatto; tuttavia, scorrendo i commi, anche quelli *ad personam*, o se si preferisce - con un'immagine più coerente con la sinistra modaiola - i commi griffati, scorrendo l'impianto complessivo di questa manovra finanziaria si ha la sensazione di trovarsi di fronte ad una sostanziale incapacità di affrontare e risolvere i grandi nodi strutturali di questo Paese. Nonostante questa manovra e, per certi aspetti, a causa di alcune misure contenute in questa manovra, si accentuano alcune questioni irrisolte: la questione salariale, la questione previdenziale, la questione della competitività e della crescita, insomma la questione complessiva della modernizzazione del Paese, sullo sfondo, appena accennata, resta la grande questione dello sviluppo del sistema Paese, attraverso la capacità di costruire condizioni di sviluppo per il Mezzogiorno. Il presidente Prodi, proprio in queste ore, ha cercato non di fare autocritica, ma di segnalare errori tattici o errori di metodo. La verità è che questa finanziaria è nata all'interno della vecchia triangolazione Governo-Confindustria-sindacato, è nata all'interno del vecchio schema concertativo. Non per un errore, ma per una scelta che rappresenta quasi un fattore, un elemento costituivo del centro-sinistra. Non la superficialità dovuta alla confusione della finanziaria, ma l'espressione di un'alleanza politico-sociale: non a caso, nella finanziaria si ritrovano alcuni punti e alcune questioni che sono tutte interne a quell' alleanza di interessi, a quel vecchio schema concertativo, incapace di leggere la realtà produttiva, associativa e rappresentativa vera del Paese. Da ciò si determina questa sorta di ossimoro della concertazione escludente che riguarda pochi ed emargina molti, come puntualmente è accaduto in questi mesi. Lo dico perché vi sono alcune questioni centrali, fondamentali, in questa finanziaria, che sono tutte interne a questa logica e a questa impostazione, a partire da quella che il Governo sottolinea con più enfasi, cioè la cosiddetta riduzione del cuneo fiscale, che viene fatta passare come un provvedimento fondamentale e strategico per la competitività del sistema produttivo. In realtà si tratta di una scelta di corto respiro, di corto respiro, che ripropone sostanzialmente, nell'epoca dell'euro e della moneta unica, ciò che accadeva nella prima Repubblica attraverso le cosiddette svalutazioni competitive, che erano sostanzialmente manovre emergenziali per restituire competitività a breve al sistema produttivo, senza affrontare le grandi questioni e i grandi nodi strutturali.

la vicenda emblematica e paradigmatica del trattamento di fine rapporto. Ho sentito parlare il senatore Caprili, con un qualche ottimismo, di consenso differito a proposito delle riflessioni del Presidente del Consiglio. Nell'attesa del consenso differito, intanto si è messo mano al salario differito dei lavoratori. Lo si è fatto attraverso un'operazione dirigista, un' operazione autoritaria,

durante gli anni del Governo Berlusconi, tra Governo e parti sociali per arrivare a soluzioni partecipate e condivise sul trattamento di fine rapporto e sulla partenza della previdenza integrativa e dei fondi pensione in maniera massiccia. Allora, attraverso la discussione, attraverso il confronto, attraverso lo scontro si è arrivati ad un punto di intesa che ha riguardato 23 organizzazioni, ABI compresa,

per consentire una scelta motivata al lavoratore. Il Governo è intervenuto in questo processo, ha stracciato l'avviso comune, ha determinato le condizioni per la scelta del trasferimento del TFR all' INPS compiendo un' operazione non di cosmesi contabile o di finanza creativa, ma di finanza truffaldina,

dai lavoratori. Mirafiori non è un incidente di percorso. Mirafiori è la consapevolezza di Cipputi di un sindacato subalterno nei confronti del Governo amico. amico. Se avessimo fatto noi, se l'avesse fatta il Governo Berlusconi quell'irruzione autoritaria sul TFR dei lavoratori, il sindacato avrebbe riempito le piazze e le fabbriche di scioperi e di assemblee. In questo caso, invece, non ha mosso un dito: ha blaterato e balbettato di autonomia e si è mosso in funzione subalterna, perché la finanziaria sta dentro quello schema, sta dentro quell'alleanza d'interessi, sta in quel meccanismo triangolare di cui parlavo all'inizio. una vicenda emblematica, che crea questa situazione paradossale. Come si fa a dire: abbiamo anticipato al 2007 la partenza dei fondi pensione perché li riteniamo, com'è ovvio, strategici rispetto al secondo pilastro previdenziale e capaci di accompagnare le nuove generazioni verso la pensione del futuro in maniera più decorosa, più decente, più adeguata, se poi si decide di mandare il TFR al fondo presso l'INPS, e si calcola di costituire un fondo pari a 6 miliardi di euro, il che significa, di fatto, tagliare le gambe alla partenza dei fondi pensione? Per questa strada, dopo avere impostato una manovra che non mette al centro il lavoro, anzi che divide lavoro e mondo produttivo, lavoro

In questa manovra c'è un altro grande assente, che pure è stato un elemento fondamentale della campagna elettorale del centro-sinistra: la centralità dello sviluppo del Mezzogiorno, del Mezzogiorno, che in una finanziaria in cui il Fondo per le aree sottoutilizzate, dopo essere stato saccheggiato dal dibattito sulla finanziaria alla Camera, si ritrova oggi in una dimensione addirittura

La verità è che questa finanziaria è come il centro-sinistra italiano: un misto di dirigismo, di centralismo, di assistenzialismo, di clientelismo, di capitalismo assistito o, più nobilmente, di radicalismo, di antagonismo, di moralismo, di sociologismo, di relativismo e di cinismo. Né massimalismo, né riformismo. Il prodismo è un *mix* originale di zapaterismo, di blairismo, di dalemismo e di mastellismo. Un fenomeno surreale, come è surreale questa finanziaria.

testo di 1.367 commi finalizzato solo a determinare il passaggio, sotto la Presidenza, del voto favorevole di qualche parlamentare, di qualche ex amministratore comunale o, ancora,

il popolo non è più con voi. E mi fa sorridere il presidente Prodi quando parla dei fischi organizzati dal centro-destra, quando gli amici dell'opposizione ci hanno spiegato che è un malessere generale del Paese.

Signor Presidente, le condizioni in cui si svolge il nostro dibattito sono certamente anomale: un grande provvedimento, costituito da un solo articolo con più di 1.300 commi, unito a un *iter* parlamentare monco. Né la Commissione bilancio di Montecitorio né quella del Senato hanno concluso i loro lavori esaminando compiutamente il testo e in entrambi i rami del Parlamento il voto finale avverrà con l'apposizione della questione di fiducia. Le nostre ultime giornate di lavoro sono state avvelenate dalle polemiche su questioni che poco hanno a che fare con la politica economica e con la sessione di bilancio. Credo che dobbiamo interrogarci sugli errori commessi. Lo faccio prima di tutto io, che avrei dovuto svolgere l'intervento iniziale del nostro dibattito come relatore sul provvedimento; ero consapevole di quel ruolo e ho lavorato con molto impegno in queste settimane. Purtroppo, le cose che avrei detto e i ragionamenti che avreifatto appaiono improvvisamente lontani, travolti da una polemica che poco ha a che fare con la legge finanziaria e alla cui origine continuo a vedere soltanto la confusione delle ultime giornate e l'affanno di un lavoro smisurato, che ha concentrato in poche ore la redazione di un testo impegnativo che avrebbe dovuto essere il frutto di lunghi giorni di discussione in Commissione. Ci sono stati errori anche del Governo. La finanziaria nasce troppo grande fin da settembre. Nella mole di 236 articoli che si occupano di tutto è difficile cogliere il filo conduttore di una strategia, le cose veramente importanti, quei muri maestri di cui ha più volte parlato il Ministro dell'economia. Anche la maggioranza parlamentare, alla Camera e al Senato, non sempre è stata all'altezza di un progetto per il Paese, che chiede di guardare alle grandi scelte e colloca in secondo piano le tante, dignitose questioni dei territori, delle categorie, degli interessi. Abbiamo commesso degli errori, dunque, e non mi sembra giusto far finta di niente, pensare che tutto possa essere rifatto come prima. Questa constatazione, questo riconoscimento trasparente non è la premessa di una resa; anzi, è la condizione per poter affermare con più forza le nostre ragioni e per guardare con determinazione alla strada che abbiamo davanti. Dall'inizio degli anni novanta l'Italia ha un problema: non riesce a crescere, a diventare più ricca. Se non si crea ricchezza, manca il lavoro, si abbassa il livello dei servizi, si deteriorano le infrastrutture materiali; ci rimettono tutti, soprattutto i più poveri. Di fronte a questa grande sfida, negli ultimi cinque anni il centro-destra ha registrato la sua sconfitta più dura. La crescita zero, che ha caratterizzato tutti i primi anni 2000, è stata lo specchio di un'economia che non riesce a risolvere i suoi problemi strutturali e scivola verso il basso nella competizione internazionale. Certo, non è stata soltanto colpa dei Governi. Ma come abbiamo detto più volte, nei cinque anni passati è stata sbagliata la strategia di politica economica, nell'illusione che bastasse una politica basata sul rafforzamento della domanda, sulla riduzione delle tasse per risolvere il problema della crescita.

che non mi interessa, ma per fissare il punto dal quale siamo partiti e per rivendicare al disegno di legge finanziaria che stiamo discutendo, pur con i suoi limiti, la decisione di affrontare il problema che ho poc'anzi enunciato: invertire la tendenza negativa dell'economia italiana, caratterizzata da bassa crescita, calo della produttività e riduzione della capacità competitiva. Vanno in tale direzione gli interventi più importanti della manovra. La riduzione del cuneo fiscale è molto importante per le imprese perché consente di ridurre il costo del lavoro, di operare scelte a favore dell'occupazione stabile,

produttivo; una strategia di rilancio della politica industriale che individua la strada per fare finalmente delle scelte in quei settori che caratterizzano un'industria capace di guardare al futuro, al futuro, che cerca nelle cose nuove, nelle tecnologie e nelle produzioni in grado di affrontare la competitività internazionale una nuova via per continuare a crescere e per risolvere i problemi strutturali di un impianto produttivo caratterizzato da una specializzazione troppo volta al passato e al tradizionale.

Questa finanziaria è stata migliorata nelle Aule del Parlamento, anche al Senato nonostante le difficoltà che abbiamo conosciuto: le norme in materia di successione delle imprese, la rivisitazione degli studi di settore, la ridefinizione di una normativa in materia di enti locali, la rottamazione delle auto Euro 0 ed Euro 1, 1, l'individuazione, nel tema del rapporto tra il contribuente ed il fisco, di un fisco capace di restituire ai cittadini il frutto di una strategia di emersione del sommerso e dell'evasione fiscale sono tutti elementi che hanno caratterizzato il dibattito al Senato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è difficile intervenire in questo momento: avevo preparato un intervento, soprattutto in materia di sanità, ma avendo ascoltato tanti colleghi non posso esimermi

non c'è un intervento in cui non vi sia un'amarezza e una critica al Governo. Solo qualche minuto fa i giornali hanno riportato gli interventi dei giorni scorsi e di ieri dei *leader* stessi della sinistra, che in maniera elegante hanno

centro-destra di organizzare le schiere, come facevate voi, di persone che protestano, anche perché sapete benissimo che abbiamo un elettorato che ha un grande difetto: delega e, soprattutto, non ha quei fondi per poter organizzare le manifestazioni. Noi - che, lo scorso sabato, abbiamo aiutato tutti coloro che intendevano manifestare la loro rabbia nei confronti di questa finanziaria a Roma - sappiamo benissimo quali sono state le cifre

su un altro aspetto, cogliendo l'occasione di avere qui presente un grande Ministro e un grande amico (ma, ahimè, rappresentante di questo Governo): mi riferisco all'onorevole Fioroni,

a quei talassemici e a tutti quei giovani che sono stati infettati, a seguito dell'utilizzo di sangue non giustamente verificato da parte dello Stato, con virus assai pericolosi e dannosi

deriso quel Governo, l'avete accusato di non aver realizzato una grande opera, perché, tutto sommato, esistono ancora molti di questi giovani e di queste famiglie ed è un'ingiustizia che non siano stati risarciti. Allora, siete andati nelle loro Regioni a fargli

per poi non fare niente! Non vi è infatti un euro a disposizione per risarcire questa grande ingiustizia, che fa parte, a mio avviso, della coscienza di tutti noi. Vorrei sapere se il senatore Morgando - che se n'è andato - sarà ancora orgoglioso di fronte a questi signori, dopo aver affermato, poc'anzi, di essere orgoglioso

Pensate che si è deciso di ignorare tutto ciò che veniva chiesto dalla Sardegna, cioè il saldo di un debito ventennale dello Stato verso la Regione, che spostò migliaia e migliaia di sardi pagati dai sindacati e dalla Regione per venire qui a manifestare. In

Ebbene, in cambio della distribuzione in 25 anni di questi oneri e di una modifica nel 2010 della lettura dell'IVA, guarda caso, i nostri nobili rappresentanti del centro-sinistra decidono che dall'anno prossimo tutta la sanità verrà pagata dalla Regione sarda, tutti i trasporti! Immaginate: un'isola che vive di trasporti, che vive del trasporto aereo e del trasporto locale che non dico essere quasi da Paesi sottosviluppati, perché non lo è, ma credetemi, in Italia rappresenta uno dei trasporti più deficitari che ci sia e quindi ha necessità di investimenti. E tutto questo su chi va a pesare? Solo sulla Regione Sardegna. Naturalmente si dice che ci rifaremo con le tasse

non chi ha veramente i soldi, ma la classe media produttiva, i piccoli artigiani, quelle persone che, mettendo da parte alcune risorse e cercando di metterle da parte per i loro figli (per poi pagare ulteriormente tasse su quello che ai loro figli daranno), si sono

drasticamente tutta l'Italia e in particolar modo il Mezzogiorno. Infatti, se andate a leggere veramente i dati, se andate a rivedere il vostro DPEF, i vostri dati, i dati che ci avete dato voi quest'estate, vedrete che il Mezzogiorno riceve meno fondi

quindi io non posso trascurare il grave danno che stiamo per affrontare. Ma soprattutto, permettetemi ancora una volta, abbiate almeno la delicatezza di non insistere nel dire che è una grande finanziaria, che non c'è niente di male se ha quasi 1.400 commi. Vorrei sapere dov'è il il vostro senatore Ciampi, che nella scorsa legislatura, perché erano 600 i capitoli di spesa, non voleva firmare la finanziaria. Dov'è? La voterà questa finanziaria che ha quasi 1.400 commi? una finanziaria per la quale avete chiesto la fiducia alla Camera, dopo di che avete detto: faremo delle modifiche al Senato. L'avete totalmente cambiata! È un film nuovo, è totalmente modificato, e voi stessi ridevate perché ogni giorno cambiava qualcosa. E allora, vi chiedo: sicuramente un metro di misura differente, ma come fate ad essere orgogliosi? Come fate ancora ad avere questa sfacciataggine? Onestamente ho grande ammirazione per voi,

tutti coloro che sono intervenuti hanno detto che creerà problemi alla propria categoria, di cui tutti hanno parlato in generale tessendone gli elogi, ma, appena sono entrati nello specifico che conoscevano meglio, hanno fatto una critica. E allora, se sommiamo tutti gli specifici, è una schifezza quella che state facendo! State realizzando una finanziaria che di fatto non taglia gli sprechi, che sta semplicemente cercando di accontentare chi vi ha permesso di arrivare al potere! Il vostro *leader* della Sardegna l'altro giorno, in maniera un po' spudorata, rivolgendosi alla minoranza (ma credo che fosse la maggioranza), ha detto: cari signori, voi dovete ringraziare che ci sono io, altrimenti sareste senza stipendio. Se avete coraggio, fate una mozione di sfiducia, dimettetevi, lo chiedo anche a voi al Senato! Se voi veramente credete che questa finanziaria sia una schifezza, come fate a votarla? Abbiate il coraggio di ribellarvi, non cercate di nascondervi dietro questa terminologia da quattro soldi per mascherare la vostra insoddisfazione e mantenervi la poltrona!

*(FI)*. Signor Presidente, i toni di questa polemica, che non è solo polemica ma è la rappresentazione anche in quest'Aula di tutta la nostra contrarietà a questo provvedimento, Colgo l'occasione, intervenendo dopo il senatore Morgando che come me fa parte della Commissione bilancio che ha esaminato questo provvedimento, per ringraziarlo per il paziente lavoro da lui svolto in qualità di relatore ogni giorno di questi lunghi giorni in cui la Commissione bilancio ha tentato di esaminare tutto il corposissimo provvedimento proposto dal Governo, provvedimento proposto dal Governo, nel tentativo (il relatore, ma anche gli altri membri della Commissione bilancio e della maggioranza) di ricomprendere tutte le contraddizioni e tutte le difficoltà che ogni giorno il provvedimento faceva sorgere all'interno della maggioranza. al presidente Morando va il ringraziamento del mio Gruppo, in Commissione bilancio, e dell'intero gruppo di Forza Italia per la grande attenzione posta alla forma e per il rigore che egli ha voluto garantire all'interno della Commissione bilancio nell'esaminare provvedimenti governativi spesso astrusi, spesso non poggiati su garanzie certe di copertura finanziaria che egli è riuscito a far modificare. Il collega Vegas intervenendo ieri ha ben sintetizzato la vera domanda che si pone chi guarda con un po' di attenzione a questo provvedimento. La domanda è: perché si è voluto portare in fondo una finanziaria così pesante, così dolorosa per il Paese, dal costo sociale così alto, e che tanto è costato a questa maggioranza in termini di consenso? Quel consenso differito al quale poc'anzi il collega Viespoli è un problema che vi riguarda, perché immagino voi abbiate piena coscienza che il Paese non apprezza ma, al contrario, si contrappone a questa vostra scelta economica.

perché gli altri 18 miliardi servono a finanziare scelte discrezionali di politica economica, alcune delle quali già indicate dal senatore Morgando. Si tratta di un insieme di misure definite con il termine equivoco di «politiche a sostegno dello sviluppo» tra le quali rientrano sia il taglio del cuneo fiscale che semplici iniziative di spesa (a volte anche modeste) indicate chiaramente da questo Governo, come il rifinanziamento dei cantieri di Ferrovie il rinnovo del contratto del pubblico impiego, in modo particolare, nuovi finanziamenti alle Poste, la missione in Libano, nonché dotazioni a vari fondi pubblici a disposizione dei singoli Ministeri (come il fondo infrastrutture, il fondo per la famiglia e quello dell'occupazione). realizzare tutto ciò il Governo utilizza misure di finanza, cosiddetta, creativa, la quale può giustificarsi se le coperture finanziarie esistono veramente, ma non si giustifica,

Lo sbilanciamento a favore delle entrate non è quindi leggero: si va ben oltre il 50 per cento e, solo in rari casi, è prevista l'attivazione di meccanismi virtuosi che porteranno a risparmi crescenti nei prossimi anni.

di finanziare le infrastrutture con i soldi del TFR, dunque ciascun lavoratore differisce il proprio salario per finanziare le infrastrutture che voi dite di voler Ma quella parte di trattamento di fine al rapporto accumulato ogni anno dai lavoratori, giovani e meno giovani, e non dirottato ai fondi pensione è già una scommessa persa, perché si tratta, in altre parole, di un prestito forzoso, per finanziarie spese infrastrutturali, ottenuto trasferendo dalle imprese allo Stato un debito nei confronti dei lavoratori dipendenti, che non eserciteranno l'opzione di trasferire il TFR ai fondi pensione. Questa misura, quindi, rischia di diventare la pietra tombale sulla speranza di creare fondi pensione in Italia perché indurrà questo Governo e quelli successivi a ostacolare in tutti i modi i flussi verso i fondi pensione. Significa meno entrate per lo Stato. Dunque è un'operazione che va a svantaggio dei lavoratori più giovani, quelli che hanno maggiormente bisogno di previdenza integrativa per garantirsi un reddito adeguato, quando andranno in pensione. Voi, quindi, scommettete sul fatto che i lavoratori dirottino verso l'INPS il loro TFR; e, se questo non avverrà, come potrete finanziare le infrastrutture? Se questo, invece, avverrà, forse finanzierete le infrastrutture e i lavoratori, sopratutto quelli più giovani, non avranno la possibilità di vedersi Noi siamo qui in Aula, oggi, a rappresentare tutto il nostro dissenso, contro questo Governo che vuole saccheggiare i nostri redditi e i nostri risparmi, impoverendo il Paese e impedendo la crescita economica. Noi siamo a rappresentare non solo l'amarezza, ma lo sdegno degli italiani, perché questo è un Governo contro: contro l'economia, contro il lavoro, contro il risparmio, contro la proprietà, contro l'impresa, contro le professioni, contro gli artigiani, contro il commercio, contro la scuola, contro l'università, contro la ricerca e contro la famiglia, che è sempre più gravata di maggiori tasse. È un Governo contro i cittadini, quindi, che ha diviso gli italiani, che divide l'Italia, che instilla nelle vene del nostro Paese l'invidia sociale, invece di promuovere la concordia e la solidarietà tra le classi. Siamo in quest'Aula per protestare contro una finanziaria che si riduce a una sola voce: più tasse per tutti. Più tasse sugli stipendi, più tasse sui BOT e sui CCT, più tasse sulla salute, più tasse sulla casa, più tasse sulle imprese. Avete gridato: «Anche i ricchi piangano!». Ma li abbiamo visti i ricchi a cui pensate voi, manifestavano il 2 dicembre in questa città: erano artigiani, accanto ai piccoli e medi imprenditori; ricercatori, i precari dell'università accanto ai rettori; i professionisti, i commercianti; i pensionati di ogni categoria, anche quelli che hanno sfilato sfilato qualche anno fa con le bandiere rosse della CGIL; il popolo dei piccoli risparmiatori, dei BOT della prima casa conquistata con una vita di sacrifici; i cittadini che vivono di uno stipendio appena dignitoso. Siete riusciti persino a spingere in piazza per la prima volta le forze dell'ordine e le Forze armate, alle quali invece tutta l'Italia deve riconoscenza. Sarebbero questi i ricchi che devono piangere? Per questa sinistra e per questo Governo sì.

negli ultimi trent'anni è la prima volta che una legge finanziaria arriva in Aula senza che siano conclusi i lavori di Commissione e quindi senza relatore. La sinistra, illudendosi di convincere i cittadini, incolpa la CdL per lo sconsiderato ostruzionismo. Ma vi rassicuro: ai cittadini non interessa la scenografia del Palazzo. I cittadini vogliono vivere e lavorare senza l'ingerenza dello Stato. Da sinistra e da destra si grida (a sinistra si mugugna, per ora) che questa gestione è antidemocratica. Gli stessi membri del Governo (sempre mugugnando) si scambiano accuse di eccessivo protagonismo e di incompetenza. I senatori ammettono di non capire né i contenuti, né tantomeno la logica economica e politica di questa interminabile lista di commi. Le agenzie lanciano le prime avvisaglie di un imminente rimpasto di Governo. Tra i Democratici di Sinistra il disagio lievita con evidenza. E Prodi? Il vostro capo? Il genio della riscossa nazionale? Lui cosa dice? Non sono preoccupato, gli italiani, anche se sono impazziti, si adatteranno a questa mazzata per il bene supremo del Paese. Veramente belle parole. Ma non tutti la pensano così. Emma Bonino così esprimeva il suo giudizio su Prodi, presidente della Commissione Europea: cervello piatto. Il «*Financial* *Times*» scriveva: la sua presidenza è stata orrenda E ancora: è un dilettante, catapultato su una poltrona troppo grande per lui. Il «*Die* *Welt*» (tedesco): impacciato, dal linguaggio piatto, un uomo che perde spesso il filo del discorso dando l'impressione di non capire di cosa si stia parlando. Qualcuno potrebbe dire che oggi è a Roma, non più a Bruxelles, ma i maligni sostengono che, anche spostandosi a sud, le doti di un *leader* non migliorano. Tutti ammettono che questa finanziaria è la peggiore dall'avvento della Repubblica e il vostro Presidente del Consiglio, il vostro capo, si indigna perché lo fischiano, teorizzando complotti e mercimonio con bande organizzate di contestatori. Perché non prova a girovagare per i mercati (quelli che si fanno nei paesi al mattino) del Nord senza darne preavviso? In questo modo potrebbe sperimentare la spontaneità dei fischi del popolo che lui tanto sottostima. Prodi ha solo due possibilità di essere applaudito. La prima è di recarsi oltralpe e dire finalmente con chiarezza (e qualcuno quindi lo deve aiutare) quello che non osa ancora dire in Italia e cioè che il Corridoio 5 (l'alta velocità) verrà spostato al nord delle Alpi, accontentando così Francia e Germania, che da sempre vogliono eliminare la concorrenza del Nord produttivo, e accontenterà anche i suoi alleati di sinistra (*no global* di Caruso compresi), che così bloccheranno in modo definitivo lo sviluppo. La seconda, più semplice e senza trasferte all'estero, è quella di dare le dimissioni per l'evidente incapacità di governare e consentire così agli italiani di tornare velocemente al voto. Se questo Governo e questa maggioranza cadessero in fretta, potremmo sperare di risollevarci perché tra pochi mesi questo Governo e questa maggioranza ci imporranno catastrofi ben più gravi di una finanziaria seppur pessima. Le unioni di fatto, i PACS e anche il diritto di adozione per le coppie omosessuali, quindi distruggere la famiglia e omologare tutti, è il sogno di questo Governo. I permessi di soggiorno regalati ai clandestini, che così arriveranno anche da tutta l'Europa, non soltanto dall'Africa. La cittadinanza veloce agli extracomunitari per avere subito il loro voto in tutte le elezioni. La riforma delle pensioni, che aumenterà l'età pensionabile. E tutto ciò che è nelle attese spasmodiche dell'estrema sinistra, che oggi condiziona Governo e maggioranza. Non sarà un sereno Natale, il vostro, colleghi della sinistra (il centro non conta più nella vostra coalizione). Le bande di contestatori, che per Prodi sono organizzate e pagate (perché non è vero, il popolo è dalla mia parte), nel giorno in cui cadrà questo Governo si trasformeranno in vere bande, che suoneranno a festa in tutte le piazze celebrando la liberazione.

desidero illustrare brevemente perché voterò questa finanziaria insieme ai miei tre colleghi eletti nella circoscrizione estero nelle liste dell'Unione. I capitoli di spesa del Ministero degli affari esteri, direttamente riconducibili agli italiani residenti all'estero, come ad esempio l'assistenza diretta e la diffusione della lingua e cultura italiane, avevano subito nel progetto di finanziaria un taglio complessivo di circa 12 milioni di euro. Il lavoro svolto dai parlamentari dell'estero e dal Governo portarono da subito un incremento di 14 milioni di euro, che coprivano i tagli annunciati. Nel maxiemendamento, sempre con la stessa modalità di lavoro congiunto, i parlamentari della circoscrizione estero della maggioranza con il Governo hanno portato a ulteriori 10 milioni di euro di finanziamenti per i capitoli prima ricordati. D'altra parte, l'impegno dei quattro senatori dell'Unione e della maggioranza tutta, con il particolare impegno del capogruppo, Anna Finocchiaro, ha fatto sì che nel maxiemendamento siano state accolte proposte di grande rilevanza per la comunità italiana residente all'estero: un finanziamento di 7 milioni, che per il 40 per cento va a beneficio delle camere di commercio italiane all'estero e per il 60 per cento ai consorzi italiani di esportazione. È stata altresì accolta la richiesta di detrazione per carichi di famiglia per i soggetti non residenti in Italia, ma è stata anche introdotta un'importantissima innovazione che riguarda direttamente tutti i cittadini italiani residenti all'estero. Infatti, dal 1° giugno 2007, i consolati italiani dovranno rilasciare e rinnovare la carta d'identità italiana ai cittadini italiani iscritti all'AIRE alle stesse condizioni degli italiani residenti in Italia. In questa finanziaria troviamo altri elementi che interessano positivamente la comunità italiana all'estero. Per esempio, la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri. A questo punto il Governo ha deciso l'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera. Questa decisione è sicuramente un segnale positivo, ma di gran lunga insufficiente per affrontare il problema della rete consolare italiana all'estero, sulla quale tornerò più avanti. Per quanto riguarda l'internazionalizzazione realizzata da consorzi di piccole e medie imprese, la valorizzazione del marchio *made* *in Italy*, i servizi postali per l'editoria destinata alle comunità italiane all'estero, il piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, non illustro tali punti, la loro positività mi appare evidente. Sull'ultimo punto, la razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, vorrei qui ricordare che lo Stato è proprietario di un immenso capitale immobiliare all'estero, che va sì razionalizzato, come dice la finanziaria, ma va soprattutto valorizzato. In questa operazione di razionalizzazione e valorizzazione, è importante che il Governo acquisisca anche il parere dei COMITES (i comitati degli italiani all'estero eletti), non solo perché sono i rappresentanti degli italiani che vivono in quei territori, e ne conoscono dunque i bisogni, ma anche perché conoscono la realtà economica degli stessi territori. Questa consultazione mi appare importante principalmente per due motivi: in primo luogo, quello strettamente economico, legato alla conoscenza del territorio; in secondo luogo, per garantire la trasparenza degli interventi ed evitare le denunce di situazioni strane che mi stanno pervenendo in questi giorni, come, per esempio, a Nizza e a Locarno, sulle quali interverrò nelle opportune sedi. Se questi sono i punti per me positivi della finanziaria, non posso non esprimere il mio rammarico per le altre nostre proposte che non sono state accolte, come la detassazione del passaporto per gli emigrati italiani ultrasessantenni, il riconoscimento pieno del sindacato dei contrattisti impiegati nei consolati, la garanzia di interventi per la formazione professionale all'estero. Continuo a pensare che il Governo avrebbe potuto rispondere positivamente a queste richieste minime, alcune delle quali addirittura a costo zero. Solo un *deficit* di dialogo che il Governo ha con la propria maggioranza può spiegare questa scelta. È nell'interesse del Paese che questo *deficit* si colmi al più presto. Gli elementi positivi della finanziaria non ridimensionano il bisogno di riforme profonde e urgenti che la comunità italiana nel mondo aspetta da questo Governo e da questo Parlamento. alla riforma del Ministero degli affari esteri. Su questo punto non si tratta di immaginare una semplice ristrutturazione, sono necessarie due componenti: innanzi tutto, una presa di coscienza di tutto il mondo politico che non si realizza una politica estera forte, capace di riscuotere consenso e il rispetto della comunità internazionale, se non si aumentano sostanzialmente le risorse economiche del Ministero degli affari esteri; secondariamente, non si ristruttura una rete consolare ridotta in condizioni miserevoli, ma bisogna ridefinire nuove regole, nuove modalità di funzionamento e di gestione del personale. Tutto ciò sarà possibile se ci sarà un largo consenso politico capace di sbloccare vecchie incrostazioni amministrative e anche, a volte, ingiustificati privilegi. Una riforma profonda, rapida e innovativa dei servizi consolari e diplomatici nel mondo porterà sicuramente ad un risparmio e ad un aumento dell'efficienza della rete consolare e diplomatica, che migliorerà i servizi sia per gli italiani residenti all'estero, sia per l'Italia in generale. Urge anche la riforma della legge n. 153 per la diffusione della lingua e cultura italiane. Alla luce della presenza dei parlamentari italiani eletti nella Circoscrizione estero, vanno urgentemente riformati il Consiglio generale degli italiani all'estero, il Comitato degli italiani all'estero e, la legge elettorale per la Circoscrizione estero. Anche la fiscalità italiana per gli italiani all'estero va ripensata: l'ICI, la tassa sui rifiuti, la tassa sui passaporti, eccetera. L'informazione degli italiani all'estero va riprogettata con la riforma dell'editoria, della diffusione della RAI in Europa, di «RAI *International*», e dell'informazione di ritorno degli italiani all'estero per l'Italia. In questo quadro vi è la necessità della risoluzione imminente dei problemi di assistenza sociale dei nostri concittadini che purtroppo all'estero non hanno trovato tutti fortuna e che nella loro vecchiaia vivono sotto la soglia della povertà, soprattutto in America latina. Non entro nel merito di queste urgenze, ma voglio dire al Governo con estrema chiarezza che su questi punti non accetteremo di perdere del tempo in indefiniti rinvii, né intendiamo avallare semplicemente decisioni prese senza la dovuta consultazione dei vari livelli di rappresentanza istituzionale degli italiani all'estero (COMITES, CGIE e parlamentari, nonché del mondo associativo), ma soprattutto non accetteremo di affrontare queste riforme con il *deficit* di confronto e di dialogo che abbiamo vissuto in questi primi mesi di legislatura. Presidente, colleghe e colleghi, mi avvio a concludere il mio intervento dando alcune informazioni che illustrano l'apporto degli italiani all'estero all'economia italiana. Mi rendo conto che finora il mio intervento ha dato l'impressione che gli italiani all'estero abbiano solo delle richieste da avanzare all'Italia. Voglio qui brevemente illustrare come la frase: «Gli italiani all'estero sono una risorsa» non è uno *slogan*, bensì una realtà. Nel 1998 il contributo degli italiani all'estero alla bilancia commerciale italiana ammontava a circa 56 miliardi di euro a fronte dei 500 milioni di euro, elargiti dal Governo per i vari capitoli del Ministero degli affari esteri. I contributi spaziano dalle rimesse agli investimenti, dal turismo di ritorno al mercato di beni e servizi (macchinari, generi alimentari, eccetera). Le rimesse dirette, pari a 2 miliardi di euro nel 1997, avrebbero potuto sicuramente essere più cospicue se ci fosse stata una politica valutaria diretta ad incentivare gli investimenti. «L'italianità» ha favorito la creazione all'estero di imprese d'importazione di prodotti e macchinari italiani. Secondo una stima del 2000 un terzo del volume delle esportazioni italiane è da attribuirsi alla presenza della rete delle comunità italiane all'estero. E le statistiche lo dimostrano: in molti Paesi, dove la nostra presenza è particolarmente consistente, il saldo fra importazioni ed esportazioni è attivo a favore dell'Italia (fonte del Consiglio generale degli italiani all'estero del 2000). Presidente, colleghe e colleghi, per queste considerazioni, sono convinto che questa finanziaria - al di là del percorso difficile, degli errori di comunicazione e quant'altro abbia dovuto e dovrà ancora affrontare - sarà in grado di far fronte ai bisogni del Paese perché porta in sé le prime risposte ai problemi che da anni frenano la nostra Italia. Una caratteristica di questa finanziaria, a mio modo di vedere, che la contraddistingue dalle ultime, è che quella attuale è ispirata da una volontà politica di interventi veri, concreti e non da una politica di mere dichiarazioni e di facciata.

Ed è per questo che tutto il lavoro positivo che abbiamo fatto per migliorare la finanziaria è un giusto e buon lavoro che non può essere sminuito e svalorizzato da sterili attacchi strumentali ad effetti mediatici. Ai detrattori di questa finanziaria, che sicuramente non è perfetta, do volentieri appuntamento fra qualche mese e credo che ci rincontreremo in un ben altro clima. Annuncio così il mio voto favorevole alla finanziaria 2007 e la mia fiducia al Governo.

Signor Presidente, colleghi e colleghe, mentre ci accingiamo a varare questa finanziaria, a concludere il primo anno della legislatura e mentre ci attrezziamo al lavoro dei prossimi anni non possiamo eludere una domanda, per inquietante che sia: perché c'è e da dove nasce il calo di consensi nei confronti di questo Governo e di questa maggioranza? un canale di «Sky», il Presidente del Consiglio ha fornito una risposta solo in parte convincente. Ha detto Prodi che nella società italiana sono presenti, operanti e forti forti molte pulsioni particolaristiche, che c'è una difficoltà ad accontentare tutti: questo è il verbo preciso che ha usato il nostro Presidente del Consiglio.

e dalla cultura imposta dal quinquennio berlusconiano. Viviamo allo stesso modo una fase lunga di crisi della coesione sociale

ma credo che ciò non sia esaustivo e non dia conto della complessità della situazione. Credo ad esempio che non sia possibile, non sia corretto, ridurre la protesta dei rettori, pur nella forma violenta e perfino un po' infantile con la quale si esprime, semplicemente a una pulsione corporativa. Credo non sia giusto ridurre l'insoddisfazione diffusa nel mondo del lavoro, anche rispetto a provvedimenti come quello sul TFR, a qualcosa di egoistico. credo che la protesta, il dissenso esplicito di molte aree del movimento e dei movimenti che si collocano nettamente a sinistra, non possano essere liquidati semplicemente come un'insorgenza corporativa. Allora il nostro problema è anzitutto quello di capire, per adeguare la nostra iniziativa e la nostra prospettiva anche alla capacità di risposta che dobbiamo rapidamente mettere in campo. Propongo qui, nel breve tempo che c'è, soltanto due spunti analitici. Appunto per capire da dove nasce questo disagio, credo sia corretto ritornare ritornare allo spirito delle elezioni del 9 e 10 aprile. I milioni di persone, la maggioranza che ‑ nonostante tutto, e i pochi voti di margine ‑ ha scelto l'Unione, lo ha fatto con una grande, forte, intensa richiesta di mutamento. Lo ha fatto investendo nel nuovo Governo, e nel mutamento che voleva fosse messo in campo, una grandissima speranza e una fortissima attesa. Ecco, questo elemento non va dimenticato, perché, appunto, più grande è l'attesa, più forti sono le domande, più forti sono le esigenze e più grande può essere oggi la delusione. L'altro giorno, incontrando una delegazione di rappresentanti sindacali, mi ha molto colpito l'affermazione di un dirigente della CGIL che esprimeva il malessere di una piccola categoria, di un pezzo dei lavoratori ATA della scuola. Diceva quel sindacalista: noi non siamo qui a negoziare, ad aprire una trattativa con questo Governo, noi

trovare naturale e normale che dal Governo Berlusconi quei diritti fossero stati ampiamente disattesi e anzi calpestati, ma trovava intollerabile l'idea che questa

Questo risarcimento, questo riconoscimento dei diritti è un punto fortissimo delle richieste del popolo dell'Unione. Aggiungo solo una piccola conclusione, che è anche il secondo elemento analitico che volevo proporre alla nostra riflessione. Prodi ha ricordato il 1996; anche a me è venuto in mente che nel 1996 fu proposta una tassa per l'ingresso in Europa: su questa tassa

perché era un obiettivo chiaro e dentro un obiettivo chiaro credo molti siano pronti anche a sacrificare i propri particolarismi. Credo che il nostro Governo, la nostra maggioranza abbia bisogno urgente non di altre fasi, non di «fasi due», non di «fasi tre» e nemmeno di «fasi uno», ma di rimettere al centro un nucleo forte della propria iniziativa politica.

Signor Presidente, signor Ministro (le do il benvenuto: è la prima volta che ella viene qui al Senato, nonostante le tante difficoltà che ha visto questa Assemblea), signori senatori, è davvero questa una brutta finanziaria, una finanziaria da bocciare, stigmatizzata dalle società di *rating*, criticata dai giornali internazionali, dagli economisti che contano, non soltanto del centro-destra, ma anche del centro-sinistra, dal governatore

La sinistra dice che lo fa in nome di un principio di equità sociale, attraverso una redistribuzione del reddito che toglie ai ricchi per dare ai poveri, ma è un'operazione Robin Hood bugiarda, perché per questa finanziaria bastano 1.350 euro al mese in busta paga (la busta paga di un operaio specializzato) per essere considerato un ricco destinato a piangere; e hanno pianto, una settimana fa, gli operai di Mirafiori. Coloro che in teoria dovrebbero essere i maggiori beneficiari della cosiddetta redistribuzione del reddito hanno criticato duramente questo Governo, ma l'equità sociale, signor Ministro, non si realizza togliendo ai cosiddetti ricchi, ma aiutando i poveri. E come li hanno aiutati? Bastonandoli tutti indistintamente, mettendo tasse sulla famiglia, mettendo tasse sulla casa, sul pronto soccorso, sui risparmi; hanno ripristinato anche la tassa di successione, dicono per grandi patrimoni, ma, con la rivalutazione degli estimi catastali e con la rivalutazione degli immobili nel tempo, hanno colpito i piccoli patrimoni, che hanno costituito il sacrificio di tanti anni di famiglie che vogliono lasciare ai figli il segno del proprio lavoro. Quindi tasse, soltanto tasse; una volta ci insegnavano all'università che le tasse erano il corrispettivo di un servizio, ma quali sono i servizi in più che sono stati dati a fronte delle tasse? Niente, anzi li hanno tolti, i servizi, se è vero che hanno tolto risorse anche agli enti locali e questo significa privare i cittadini di servizi fondamentali, come l'assistenza agli anziani, i servizi sociali, i buoni mensa, gli asili nido. Chi farà le spese di tutto questo? Naturalmente, e sempre, le persone più deboli che, appunto, la sinistra diceva di volere tutelare.

Occorre fare emergere il lavoro nero, il sommerso, bisogna far pagare le tasse a chi non le ha mai pagate, non a chi le ha sempre pagate.

Ma questo è uno Stato che non governa e non persegue un controllo virtuoso della fiscalità, che sopraffà e schiaccia i cittadini con effetti che potranno essere contrari a quelli perseguiti. Le vendite nei negozi sono diminuite, gli investimenti sono bloccati, i capitali stanno andando all'estero. L'economia è totalmente bloccata. Noi abbiamo ereditato nel 2001 un buco di 35.000 miliardi delle vecchie lire e abbiamo lasciato alla sinistra al Governo del Paese un gettito fiscale incrementato di un punto percentuale sul PIL,

futuro ai nostri giovani. È una finanziaria punitiva nei confronti del ceto medio produttivo, quel blocco economico e sociale che costituisce il tessuto sano del nostro Paese. È una finanziaria che ha provocato uno scontro sociale senza precedenti nella storia del nostro Paese. Due milioni di persone sono scese in piazza il 2 dicembre scorso per manifestare un disagio profondo. Per la prima volta, tutte le categorie economiche e sociali si sono unite nel dissenso; per la prima volta, ci sono stati scioperi importanti come quelli delle Forze dell'ordine; per la prima volta, le università, come quella di Padova, hanno decretato la disobbedienza fiscale. Non era mai successo. successo. Queste categorie nella finanziaria non sono state neppure interpellate nella elaborazione dei vari emendamenti e articoli, alla faccia del tanto sbandierato criterio della concertazione.

Senza contare l'aumento, del quale non si parla ma che ci sarà, attraverso la rivisitazione degli studi di settore. Noi riteniamo che più tasse significhi blocco dello sviluppo; che meno sviluppo significhi meno entrate; che meno entrate significhi più spesa

Non è la difesa di piccoli interessi o delle categorie, non è una difesa corporativa. E' la difesa di un modello di società incentrata sul cittadino

*(Misto-Pop-Udeur)*. Signor Presidente, colleghi senatori, le leggi finanziaria e di bilancio sono strumenti contabili fondamentali per la gestione delle risorse statali. Prima di qualsiasi valutazione sul merito tecnico-normativo dei provvedimenti, intendo ricordare e ribadire quanto programmato dal nostro Presidente del Consiglio all'indomani del voto alla Camera Prodi, infatti, affidandosi all'autore del provvedimento, mente eccellente dell'economia, ha ribadito la necessità di una manovra rigorosa, puntando su una finanziaria di sviluppo e di equità, non limitandosi al minimo indispensabile. La scelta è propria del buon Governo, che il saggio Tucidide avrebbe definito del «potente per dignità», cioè delle istituzioni che appaiono severe verso il popolo, senza però limitarne in alcun modo la libertà. Ma c'è un altro dato riscontrato e rimbalzato alla mia mente quale risultante degli incessanti lavori in 5a Commissione. Ancora una volta, purtroppo, ha prevalso la competizione al vero senso della politica che è, viceversa, serio confronto e scambio. Sono convinto, infatti, che nel confondersi dei periodi storici tutti abbiamo dimenticato cos'è realisticamente far politica a vantaggio del Paese. Viceversa, le mie reminiscenze ideologiche mi conducono a tempi in cui far parte delle istituzioni significava lottare per un credo politico, ma anche cercare un confronto positivo con chi era dall'altra parte. In altre parole, mi sono convinto che la massiccia incomprensione delle parti politiche attuali, il mancato dialogo tra maggioranza e opposizione è diventata norma a discapito di tutti. Una prassi che ha sembianze di un cerbero che mangia la sua coda, una sorta di girotondo distorto che non conduce a buon fine ma si dirige verso strade inopportune fatte solo di arroganza, senza scambio di idee né collaborazione. Cari colleghi, mi sono reso conto che siamo in un vortice viziato senza inizio né fine, che sarebbe bene spezzare aprendo le porte ad un contraddittorio fattivo fra le parti politiche. Probabilmente questo uovo di Colombo è la chiave per aprirci nuovamente alla vera politica e percorrere una strada di condivisioni più che di sfide senza concretezze. Perdonatemi questa premessa, che può sembrare digressione, ma ci tenevo ad esortare una pausa di riflessione affinché si possa sperare per il futuro di agire con senso costruttivo per il Paese. Certamente, non nego che mettere la fiducia alla manovra finanziaria, oggi come oggi, era indispensabile sia per ragioni di tempo che per mancanza di collaborazione e di intesa tra noi e l'opposizione, ma ciò che intendo sostenere è che occorre è che occorre dare ai cittadini un'informazione giusta sulle logiche della manovra. Questa maggioranza non si nasconde dietro l'insuccesso del precedente Governo, ma intende andare oltre, anche a costo di approvare un provvedimento risultato impopolare ad una larga parte del nostro Paese. D'altro canto, lo stesso Prodi ammette con coscienza che si capirà il senso e il contenuto della nostra azione e si perdoneranno anche i nostri errori tattici; come forza politica di coalizione siamo consapevoli che questo Governo riuscirà, nonostante le polemiche, ad intraprendere un percorso virtuoso. Tuttavia, avvertiamo il rischio che il facile ricorso alla fiducia può significare svilire l'azione del Governo *pro viri*, per la società. Al di là della manovra finanziaria, che pure incombe pressante nei tempi, abbiamo ben altre responsabilità e grandi progetti normativi da realizzare, per i quali si dovrà cercare giocoforza più intesa tra le parti. Si sa, si è costantemente lavorato con l'unico obiettivo di addivenire ad una legge effettivamente democratica che, anche se per alcuni versi impone dei sacrifici, dall'altra parte si prefigge di raggiungere un risultato remunerante a lungo termine per tutte le categorie sociali. Dunque, particolare menzione va rivolta ai lavori della 5a Commissione. In due settimane non abbiamo certamente evaso il compito tortuoso di analizzare e studiare approfonditamente la manovra finanziaria, suggerendo proposte migliorative del testo licenziato dalla Camera. Non si è perso tempo! Parte di queste proposte sono state inserite nel maxiemendamento redatto dall'Esecutivo che, in tal modo, non ha vanificato del tutto l'impegno profuso. Il gravoso onere di accogliere le molteplici istanze pervenute da più parti era dovere per il Senato, che mirava ad un documento organico e più fluido sulla base delle esigenze captate dalla società civile, ed è stato dovere per il Governo proseguire in tal senso. Ovviamente in sede d'analisi non sono mancati problemi, connaturati alla delicatezza del testo tecnico; comunque mai si è perso l'obiettivo primario di raggiungere un'intesa ampia e condivisa da tutti i Gruppi di maggioranza, anche quando alta è stata la divergenza nei dibattiti. Avevamo intrapreso in materia di equiparazione di diritti tra coniugi e conviventi un terreno scivoloso. La responsabilità della maggioranza e la decisione di affrontare la questione in una fase diversa da quella della sessione di bilancio hanno evitato la *debacle*. La finanziaria 2007 non poteva rappresentare un mezzo per costringere il Parlamento a forzature legislative! Non volendo entrare nel merito dei contenuti del maxiemendamento, sottolineo che tanto di buono è stato fatto, ma tanto ancora si sarebbe potuto ottenere specie per accentuare le prospettive di sviluppo e di crescita delle Regioni del meridione e quindi di tutta l'Italia. Nuovamente si è persa una buona occasione per rendere il nostro Sud volano per l'intera economia nazionale; proprio con la finanziaria, infatti, doveva affermarsi un modello di sviluppo che ponesse al centro dei propri interventi la crescita del Mezzogiorno. Colleghi senatori, perdonatemi un'ultima valutazione. Abbandoniamo, una volta e per tutte, la prassi improduttiva e ostruzionistica che vede la legge finanziaria trasformata in un immenso calderone recettivo di ogni richiesta, anche delle più singolari e totalmente avulse dal contesto finanziario. La legge finanziaria deve tornare ad essere atto normativo volto a definire un quadro chiaro e coerente delle grandezze di finanza pubblica e ad indicare gli obiettivi prioritari della politica finanziaria da perseguire. Proprio a tale scopo, noi Popolari-Udeur abbiamo presentato un disegno di legge che mira ad una ridefinizione del contenuto e delle procedure della manovra finanziaria. È impensabile lavorare per quattro mesi incessantemente su questo provvedimento e lasciare il Paese senza la rappresentatività dei due rami del Parlamento per altri problemi, anch'essi meritevoli di tanta attenzione. Occorre infatti revisionare taluni aspetti dell'attività legislativa, che condizionano la qualità della normazione e la complessiva efficacia delle risposte che il sistema istituzionale può

anzi, eccellente proposta! Tuttavia, l'intento di riformare le procedure risulterà vano se non si tornerà a fare politica. Le singole forze dovranno iniziare realmente a rappresentare, nella manovra di finanza pubblica, le proprie visioni di politica economica generale. Concludendo, signor Presidente, colleghi senatori, in buona sostanza e senza eufemismi è stato impegnativo raggiungere l'intesa ed il Governo non poteva non tenere conto dei risultati conseguiti in sede di istruttoria. Quindi, con convinzione sono qui a sottolineare che i lavori effettuati sono preludio di una legge rigorosa, la cui funzione principale sarà quella di ridare spazio all'Italia, alla sua economia, nonché quella di rilanciare il Paese nell'ottica europea. La responsabilità che accettiamo oggi è forte ed io, a nome del Gruppo Misto Popolari-Udeur, la assumo con la sicurezza

Signor Presidente, i senatori di opposizione che mi hanno preceduto non hanno mancato di segnare lo spartiacque che divide l'Aula. sopra la ringhiera che nel Senato separa la maggioranza dall'opposizione, un punto d'incontro, in questa lunga discussione, è stato pure trovato: si tratta dell'opinione condivisa porre mano, con il nuovo anno, ad una nuova normativa della legge finanziaria, che dal 1978 accompagna, integra, modifica e complica la deliberazione del bilancio dello Stato. Se si ripensa alle origini, la legge finanziaria fu istituita allo scopo di incardinare la discussione del bilancio in ordine a due princìpi: la coerenza con gli obiettivi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed il quadro di regolazione delle grandezze finanziarie complessive. Di fatto, i modi di esecuzione di quei due princìpi lasciano adito credo ogni anno ed anche quest'anno a molti elementi di discussione. È accaduto ed accade che, di anno in anno, nella proliferazione di emendamenti, la finanziaria assuma la fisionomia di un convoglio sempre più lungo, carico di una quantità di mercanzie legislative varie e variabili, che, alla fine, possono essere padroneggiate solo da pochi addetti ai lavori di Commissione; e siccome il diavolo si nasconde nei dettagli, può succedere che saltino sul convoglio in marcia anche norme di ordinamento che nella legge finanziaria non devono trovare ospitalità, come il comma sui termini di prescrizione dei danni erariali, che immagino si provvederà a rimuovere. Ieri abbiamo ricevuto il testo conclusivo: anch'io - come, immagino, tutti - ho dedicato qualche ora a decifrarlo. però, che abbiamo degli studenti in visita, devo ammettere che, se fossi sottoposto ad un interrogatorio sul contenuto dei 1.365 commi del maxiemendamento, avrei poche speranze di superare l'esame. Ho, perciò, apprezzato l'impegno annunciato dal presidente Morando, che non a caso ha trovato generale consenso, di presentare al più presto una proposta di modifica delle procedure d'esame dei documenti di bilancio. Allo stato attuale di quelle procedure, alla fine, diventa quasi inevitabile il ricorso al voto di fiducia. Il significato politico della fiducia al Governo rialza talmente la discussione rispetto alla congerie delle norme specifiche, da restarne quasi distaccato.

Vorrei, per quanto possibile, fare a meno degli atti di fede, dunque voterò la fiducia al Governo per una duplice considerazione. Anzitutto, perché la finanziaria riporta in linea i conti pubblici, raddrizzandoli rispetto alla linea del Governo precedente, che si era mangiato l'intero avanzo primario. Poi, anche perché l'indispensabile riduzione del disavanzo è la premessa di quella combinazione fra equità e crescita che sarà il successivo banco di prova per l'azione di Governo. sulle politiche per l'equità e per la crescita che intendo esporre qualche osservazione di merito nel poco tempo che ci è concesso. Signor Ministro dell'economia, si ritiene, da parte che il fine dell'equità giustifichi l'azione redistributiva dello Stato, praticata dalla leva fiscale in misura progressiva rispetto alla capacità dei contribuenti. È spiacevolmente ovvio che, quando i redditi dichiarati non corrispondono alla capacità effettiva, il presupposto dell'equità venga meno e l'aggravio delle progressività si traduca in un premio per gli evasori e in una penalizzazione dei contribuenti reali. Considero perciò rassicurante, rispetto al testo ricevuto dalla Camera, l'innovazione ora contenuta nei commi 4 e 5 che destinano le maggiori entrate, da recuperare con la lotta all'evasione, alla riduzione della pressione fiscale; anzi, fra le modifiche apportate dal Senato al testo ricevuto dalla Camera, l'impegno ad utilizzare i proventi della lotta all'evasione per la riduzione delle aliquote mi sembra il più significativo, in quanto anche la moderazione del prelievo tributario è un fattore non secondario di equità (in questo caso, dell'equità che pure deve sussistere nel rapporto fra la mano pubblica e le tasche dei cittadini). Se si considera l'equità su quel versante, presta il fianco alle discussioni (che infatti non sono mancate, anche da fonti istituzionali autorevoli) il fatto che la riduzione del disavanzo sia ottenuta unicamente con maggiori entrate, dato che le riduzioni di spesa sono inferiori alle maggiorazioni. Vero è che le maggiorazioni di spesa sono in buona parte orientate alla crescita, e tra le azioni per la crescita vorrei porre l'accento sugli investimenti in infrastrutture richiamati poco fa dal senatore Morgando, in particolare sull'arteria europea che dovrebbe (ormai temo che il condizionale sia d'obbligo) attraversare l'Italia del Nord da Torino a Trieste. Si prova un'impressione di angoscia, signor Presidente, vedendo nei giornali la carta delle grandi comunicazioni europee con il tracciato del Corridoio 6 da Parigi a Vienna in via avanzata di costruzione e, sotto le Alpi, il tracciato del Corridoio 5, da Lione a Lubiana, che tra ribellioni localiste, varianti di fantasia, conferenze tardive, è ormai a rischio di abbandono tra lo stupore della Commissione europea, la crescente freddezza dei finanziatori francesi, la coraggiosa ma sempre più disarmata difesa che il Presidente del Piemonte e il Sindaco di Torino dedicano ad un progetto essenziale se si vuole che le più produttive Regioni italiane non siano confinate ai margini della circolazione europea. è oggi in Italia, mi sia consentito dirlo, insieme alla storica questione meridionale anche una nuova questione settentrionale, non perché le carenze delle infrastrutture e le disfunzioni dello Stato siano meno gravi al Sud che nel Nord, tutt'altro; ma perché la prossimità con le aree forti d'Europa le rende più evidenti e il differenziale comparativo incide più direttamente sulla capacità di competizione del sistema produttivo sui mercati esterni. Dunque: gli investimenti in infrastrutture materiali e immateriali, che costituiscono il capitale fisso della Nazione; la correzione dei malfunzionamenti degli apparati pubblici; la liberalizzazione nelle aree dove persistono mercati chiusi: è su scommesse di questo genere che si misura la politica di crescita di cui il risanamento dei conti pubblici costituisce la premessa la premessa necessaria. Signor Presidente, la travagliata gestione della legge finanziaria è accompagnata, in quest'Aula e fuori di essa, da incertezze, aggiustamenti, timori ed anche proteste che non sarebbe giusto e neppure possibile ignorare. Ma io non credo che la qualità di una legge finanziaria vada misurata dagli applausi e dai fischi che riceve, come si fa per i tenori della Scala. Ritengo invece importante che non si smarrisca, per compiacere alle tensioni e alle pressioni, quel senso della prospettiva che infine qualifica una strategia di Governo. Conosciamo le difficoltà oggettive con cui l'esordio del Governo ha dovuto fare i conti e le non minori difficoltà che si prospettano già da domani per l'attuazione della linea che è stata autorizzata dagli elettori. Serve in questo momento una assunzione di responsabilità comune che dia sostegno e continuità ad un'opera appena cominciata. Per questa ragione, che sorpassa tutti i distinguo,

un cacciabombardiere *Joint Strike Fighter* e dieci carri armati Ariete equivalgono grosso modo alla rata annua che l'Italia dovrebbe pagare al Fondo globale contro AIDS, tubercolosi e malaria: un impegno preso proprio dal nostro Paese, dall'allora Governo Berlusconi, nel corso del Vertice G8 di Genova, nelle stesse ore nelle quali si consumava all'esterno una delle pagine più tristi e buie della nostra storia, pagine che chiedono ancora giustizia, come chiedono giustizia milioni di donne, uomini, bambini, che ogni anno vengono colpiti dall'AIDS, dalla malaria e dalla TBC. Vite prese in ostaggio dalla logica delle grandi case farmaceutiche multinazionali per le quali il diritto alla vita e alla salute è solo una quota di mercato. Resterà una macchia su questa manovra finanziaria che per altri versi sta cercando faticosamente di segnare una discontinuità rispetto al passato: il mancato impegno a versare le quote che il nostro Paese deve al Fondo globale (20 milioni di euro di arretrati per il 2005, 130 milioni ancora da pagare per il 2006 e altrettanti per il 2007) e, per contro, la conferma di uno stanziamento enorme, a nostro parere inaccettabile, di finanziamenti per nuovi sistemi d'arma tra cui proprio il *Joint Strike Fighter*. Seppure perfettibile, il Fondo rappresenta oggi il tentativo di costruire uno sportello nel quale soggetti pubblici e privati possano mettere in *pool* le loro risorse per il sostegno ad un bene pubblico globale, quello della lotta contro le pandemie. Tra i limiti quello di non aggredire alla base le cause strutturali, le carenze dei servizi sanitari, le regole spietate del commercio internazionale, gli effetti devastanti dei piani di aggiustamento strutturale e del pagamento del tuttora pesante fardello del debito estero. debito estero, il nostro Paese ha una legge all'avanguardia (la legge n. 209 del 2000) la cui applicazione ha portato e porterà all'alleggerimento del peso debitorio di molti Paesi impoveriti. Anche quell'approccio però non basta più. La questione centrale è riportare democrazia ed equità nelle trattative sulla cancellazione del debito, pensare nuovi modelli partecipati, accrescere il ruolo dei Parlamenti, riconoscere che esistono debiti illegittimi ed odiosi che i popoli hanno diritto di non pagare. Lo ha fatto di recente il Governo norvegese, dovremmo provare a farlo anche noi. Ci apprestiamo poi a discutere anche della riforma della cooperazione e smettiamola di chiamarla cooperazione allo sviluppo, iniziamo ad usare altri termini, magari solidarietà internazionale, ma non sviluppo, giacché quel paradigma meramente economicistico ha finito per impoverire ulteriormente la maggioranza del mondo. Ebbene, questa finanziaria segna un'importante inversione di tendenza rispetto al passato, allocando 650 milioni di euro l'anno per la cooperazione. E' ancora poco, ma certamente un segno di impegno per raggiungere quello 0,33 per cento del PIL che ci chiede l'Europa. Sbaglieremmo però a confinare la questione della cooperazione solo all'aspetto quantitativo. C'è bisogno di cambiare passo, filosofia, obiettivi. L'Italia ci sta provando aderendo, tra l'altro, ad un'importante iniziativa per strumenti finanziari innovativi per la lotta alla povertà, il cosiddetto Gruppo di Rio.

Concludo il mio intervento ricordando altre due scadenze importanti per il nostro Paese, che richiedono un impegno politico forte e strumenti di lavoro adeguati, quindi finanziamenti adeguati.

della Palestina all'Afghanistan, al Corno d'Africa, alla Birmania, ai diritti del popolo Saharawi. A maggio poi si terrà la prima fase della Conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare (il TNP) dove l'Italia dovrà svolgere un ruolo di primo piano per il disarmo e la pace. Questa è la politica estera vera, la politica estera etica che noi vogliamo, che continueremo a costruire qui con questa maggioranza ma anche al di fuori, con i movimenti sociali e dal basso per cercare davvero di contribuire alla realizzazione di un mondo più giusto ed equo.

lei, ministro Padoa-Schioppa, questa mattina in un'intervista a «la Repubblica» afferma che inseguire il consenso giorno per giorno è una perdizione.

della missione che i cittadini ci hanno affidato nel momento in cui sono andati alle urne esprimendo una speranza forte di cambiamento. Il nostro Governo, la nostra maggioranza rappresenta ed ha rappresentato per molto tempo agli occhi dei cittadini proprio questa speranza, questa voglia di cambiare.

Qualcuno ha ironizzato sulla cabina di regia. Io ritengo, invece, che sia stata un'esperienza importante in cui la maggioranza si è assunta le proprie responsabilità. Al Senato abbiamo tentato di rimettere sui binari giusti la finanziaria, di superare quei problemi, quei difetti di comunicazione

come alta: una sfida alta e grande, quella cioè di conciliare insieme il risanamento, le politiche di equità, le politiche sociali e, soprattutto, una nuova qualità sociale ed ambientale per lo sviluppo.

a non farci tirare per la giacchetta - come si dice - dalle spinte di conservazione. Avevamo indicato come oggi la sfida dell'innovazione

anche al settore agroalimentare dove con un lavoro collettivo abbiamo dato un segno che qualità, innovazione e possibilità di competizione possono stare insieme e rappresentare una sfida forte per per il futuro, dopo tante chiacchiere. Oggi si concretizzano una serie di provvedimenti. Sul fronte ambientale abbiamo conseguito risultati importanti che seguono quelli della Camera. Però - lo voglio dire con forza quella perdizione che porta a non voler affrontare l'innovazione, a non volersi staccare da alcuni interessi, si è materializzata anche qui. Non si è voluti andare fino in fondo, per esempio, sull'innovazione delle energie rinnovabili. Si era costruito un percorso ma qualcosa è accaduto. Un errore materiale? Bene, sfidiamo il Governo, lo dico al ministro Chiti, a fare in modo che quell'errore materiale possa essere riparato al più presto. Altrimenti dobbiamo pensare che la seduzione della conservazione ancora una volta si insinua nelle scelte del Governo. Lo voglio dire forte: se non chiudiamo la questione del CIP6 una volta per tutte, quella vergogna, quella truffa

conservazione. Riprendo di nuovo la frase del ministro Padoa-Schioppa: inseguire il consenso giorno per giorno è una perdizione. Ma è anche una perdizione inseguire il consenso solo di una parte,

La missione che ci hanno affidato i cittadini è quella di conciliare le politiche di risanamento con le politiche dei diritti e con le politiche della nuova qualità sociale e ambientale. Non sono le richieste della sinistra radicale: è una necessità oggi e di ora per spingersi avanti davvero sul fronte del rilancio economico, della sfida, che è ancora possibile, ma bisogna superare

la perdizione per seguire i consensi di altri e riprendiamo la nostra strada verso tale missione, perché a questo i cittadini ci hanno chiamato.

Tanto grande è stata l'enfasi posta dai *leader* dell'Unione, ieri, durante la campagna elettorale, sulla necessità della coesione sociale quanto grande appare oggi il diffuso dissenso di tutti i molteplici segmenti sociali nei confronti della politica economica del Governo. E questo dissenso potrebbe tradursi in caduta dei consumi, come degli investimenti privati, in forme di conflittualità per definire la distribuzione della minore ricchezza, in vari modi di fuga dalla responsabilità dei singoli, come dei gruppi sociali. Voi avete consapevolmente presentato la manovra nel segno dell'antagonismo tra classi sociali, in quanto ne avete sottolineato gli obiettivi della redistribuzione dei redditi attraverso la leva fiscale e della cosiddetta lotta all'evasione attraverso la premeditata criminalizzazione del lavoro autonomo e delle libere professioni. Il disegno teorico era tanto chiaro quanto odioso: costruire, attraverso la clava fiscale, un blocco sociale di sostegno al Governo, fatto di pubblici dipendenti, operai della grande industria sindacalizzata, *managers* superpagati delle maggiori imprese indebitate, boiardi bancari beneficiati dal crollo procurato della prima Repubblica, editori impuri perché espressione del vizioso intreccio banca-impresa. Questo disegno di divisione del Paese, emblematica rappresentazione del miscuglio di ideologismo ed opportunismo che vi caratterizza, non è riuscito perché non poteva riuscire. La odiosa separazione dei tavoli di dialogo sociale che noi avevamo unificato, la menzogna sul nostro lascito in termini di *extradeficit*, l'incapacità di selezionare le pressioni interne sulla maggiore spesa corrente, la straordinaria dimensione del maggiore prelievo fiscale, hanno determinato quella diffusa contestazione che neppure i molti amici che avete nelle burocrazie della rappresentanza hanno potuto nascondere. Il lavoro dipendente ha immediatamente avvertito come il ridisegno delle aliquote e degli scaglioni IRPEF, combinato con il passaggio dalle deduzioni alle detrazioni per carichi di famiglia, con le maggiori addizionali locali, con l'aumento della contribuzione previdenziale e con altre imposte sui consumi incomprimibili delle famiglie, è inesorabilmente destinato a ridurne il reddito disponibile. Il lavoro autonomo ha percepito il fatto che questa è la manovra ad esso più ostile in tutta la storia della Repubblica: dalla modifica unilaterale degli studi di settore, all'incremento dei contributi previdenziali nonostante l'equilibrio delle relative gestioni, al prelievo sui contratti di apprendistato, lavoro pubblico è stato da un lato gratificato con la promessa di un buon contratto - con l'eccezione delle forze dell'ordine - ma, dall'altro, penalizzato con lo scivolamento degli aumenti oltre il biennio contrattuale. Gli imprenditori piccoli e medi hanno rifiutato l'illusione ottica del minore cuneo fiscale, largamente compensato dagli altri interventi fiscali e regolatori, come il recente codice ambientale o l'annunciata controriforma del lavoro. Perfino la volontà di penalizzare le cosiddette rendite non ha tenuto conto delle stretto intreccio tra esse ed i profitti quale si manifesta con le diffuse società immobiliari generate da imprenditori industriali per dare sicurezza alla loro accumulazione e garanzie alla capacità di indebitamento. Che cosa è rimasto quindi del vostro disegno sociale? Solo la complicità di alcuni interessati banchieri e *managers* con cui vi siete emblematicamente riuniti nel giorno in cui si svolgeva a Roma la più grande manifestazione interclassista del Dopoguerra,

gli intenti di revisionare in peggio la disciplina della previdenza pubblica e la più significativa liberalizzazione già realizzata, quella del mercato del lavoro. L'avere poi bruciato le risorse del cuneo fiscale con una manovra insensibile alla competitività non consentirà alle parti sociali quella intesa sulla produttività che richiederebbe una detassazione delle componenti premiali della retribuzione in modo da incentivare i relativi accordi aziendali. La verità è che voi siete strutturalmente impossibilitati, per le caratteristiche stesse della vostra coalizione, a produrre quella coesione tra interessi sociali di cui il Paese ha bisogno per ricostruire le condizioni di uno sviluppo economico e sociale duraturo. Per questo rappresentate un Governo pericoloso per il futuro della Repubblica. Per questo faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità democratiche, qui e fuori di qui, per mandarvi a casa. *(Ulivo)*. Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, ove depurassimo il dibattito sui documenti finanziari dalle scontate ed ovvie strumentalità politiche, si riconoscerebbe che la legge finanziaria per il 2007 è orientata, in conformità con quanto stabilito dal DPEF, al rilancio della crescita economica, in un contesto di risanamento strutturale della finanza pubblica, di equità sociale e di maggiore efficienza della spesa pubblica. La manovra correttiva riduce il rapporto *deficit*-PIL al di sotto del 3 per cento, in armonia con gli impegni assunti in ambito comunitario. La restante parte della stessa è destinata a reperire risorse, riattivare programmi essenziali di spesa a favore dello sviluppo e per interventi volti a garantire le funzioni essenziali dello Stato. Tra queste, rilevanti sono quelle relative al Ministero della difesa, sulle quali mi soffermerò in questo mio breve intervento. In questo ambito, sono state individuate come priorità la riorganizzazione e la razionalizzazione della difesa, da realizzare tra l'altro mediante l'accorpamento e la ridefinizione, in chiave interforze, delle strutture e dei comandi, per realizzare economie di scala, economie di gestione e recuperare risorse per razionalizzare tutto il complesso infrastrutturale. In secondo luogo, la professionalizzazione delle Forze armate, promuovendo nel contempo l'elevazione del livello culturale e addestrativo del personale, favorendo il benessere dello stesso, con particolare riferimento ai settori previdenziali e abitativi, valorizzando il contributo della rappresentanza militare. In terzo luogo, l'ammodernamento dello strumento militare, in grado di assicurare elevata capacità di schieramento, mobilità e proiezione delle forze, anche fuori area, nonché attraverso il potenziamento della ricerca tecnologica e del sostegno allo sviluppo dell'Agenzia europea della difesa, allo scopo di armonizzare le esigenze e i requisiti operativi e militari a livello europeo. In quarto luogo, il funzionamento dello strumento militare per garantire la piena operatività in condizioni di sicurezza e per sviluppare la capacità di operare in contesti internazionali. Al fine di realizzare tali obiettivi le disponibilità totali di competenza risultano incrementate di circa 2.085,3 milioni di euro per un totale di circa 20.219,75 milioni di euro. Le spese per l'esercizio e per l'investimento sono state è vero - oggetto di notevoli riduzioni negli ultimi anni; basti ricordare che solo lo scorso anno sono stati tagliati 1.176 milioni di euro per l'esercizio, mentre per l'investimento il taglio è stato di 1.076 milioni di euro. Ma non voglio fare una cronistoria delle riduzioni delle risorse finanziarie destinate alla difesa nel periodo 2004-2006; sarebbe facile dire che coloro come il collega Ramponi - che oggi rilevano l'insufficienza di risorse, sono gli stessi che in quegli anni governavano, decidevano i tagli e sostenevano pareri positivi in Parlamento ai tagli stessi. Questo per ricordare che la situazione da cui partiamo è l'eredità lasciata dal precedente Governo. Un'eredità davvero da fiasco colossale, sia per la riduzione delle risorse destinate agli investimenti e all'esercizio, che hanno messo in crisi le Forze armate, sia per il mancato stanziamento dei fondi nella finanziaria dell'anno scorso per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2006-2007, che ha fatto slittare di un anno il rinnovo degli stessi contratti, anche se adesso, ipocritamente, l'opposizione addebita nelle piazze, in forma demagogica, questa responsabilità e questo malcontento a questo Governo quand'esso deriva dalle scelte che loro stessi hanno determinato. Ebbene, in questa finanziaria le risorse per il rinnovo dei contratti ci sono e, in aggiunta a queste, vengono stanziati ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2007 e 80 milioni di euro per l'anno 2008 per il trattamento accessorio, la cosiddetta specificità del personale delle Forze armate e dei corpi di Polizia, nonché in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale. I provvedimenti contenuti nella precedente finanziaria del Governo Berlusconi hanno abrogato con una misura odiosa le spese di cura ospedaliere e per protesi, per le infermità dovute a causa di servizio, adesso ripristinate dal comma 556 del maxiemendamento. Quella stessa finanziaria del Governo Berlusconi ha soppresso le indennità relative ai fogli di viaggio, ripristinate poi per il personale militare, ma non per quello civile. Quella stessa finanziaria del Governo Berlusconi ha deciso tagli del 10 per cento agli stanziamenti relativi alle prestazioni del lavoro straordinario. Tutto questo, i colleghi dell'opposizione lo hanno fatto l'anno scorso con un voto di fiducia, per il quale oggi fanno tanti strepiti. Chiarito questo, mi limiterò a citare solo alcuni punti qualificanti della legge finanziaria; con stanziamenti nuovi e mirati si inverte questa tendenza negativa degli ultimi anni, relativa alla riduzione delle risorse destinate alla difesa, che ha portato il rapporto tra funzione difesa e prodotto interno lordo allo 0,825 per cento, vale a dire il punto più basso in assoluto nella storia repubblicana. Cambia la procedura di individuazione dei beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa non più utili ai fini non più utili ai fini istituzionali. Tale attività compete ora direttamente al Ministero della difesa che vi provvede con decreti da emanarsi d'intesa con l'Agenzia del demanio e non più a quest'ultima di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa stesso. È stabilito il valore complessivo degli immobili da individuare ai fini della dismissione: 2 miliardi di euro nel 2007 e 2 miliardi di euro nel 2008

del fuoco. Infine sono stanziati 30 milioni di euro per reclutamenti straordinari nell'Arma dei Carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza per esigenze connesse al contrasto della criminalità e dell'economia sommersa. Da rilevare che, relativamente alle assunzioni, le amministrazioni debbono continuare ad avvalersi del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni e prioritariamente del personale 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006, ovvero degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e delle Forze armate. È anche questo un primo passo per la stabilizzazione di personale in condizioni di precariato, nel rispetto degli impegni assunti in campagna elettorale Vi sono le poi disposizioni per incrementare i benefici economici spettanti al personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2006-2007: nell'ambito delle risorse destinate a tali benefici sono specificatamente vincolati alle Forze armate e alle Forze di polizia 304 milioni di euro per il 2007, 805 milioni di euro per il 2008 e sono stanziati ulteriori 40 milioni di euro di euro per il 2007 e 80 milioni di euro per il 2008 per il trattamento accessorio, come dicevo prima, come richiesto dai COCER e dai rappresentanti dei sindacati di Polizia. Vengono rifinanziate le attività previste in favore delle imprese nazionali del settore aeronautico, autorizzando contributi quindicennali da erogare. Rinuncio a richiamare la sequenza di tali misure per dire, in conclusione, che nello che nello Stato di previsione del Ministero della difesa si istituisce un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico. Credo che anche questo contribuisca ad aiutare la ricerca nel nostro Paese. Il Fondo è iscritto con una dotazione di 1.700 milioni di euro per il 2007, di 1.550 milioni di euro

Un ulteriore fondo di 50 milioni di euro è stato stanziato per la bonifica delle aree militari interessate dalla presenza di poligoni militari di tiro, per la ristrutturazione e l'adeguamento degli arsenali e l'ammodernamento del parco autovetture dell'Arma dei Carabinieri. Per il Corpo delle Capitanerie di porto sono stati stanziati 7 milioni di euro per il potenziamento della componente aeronavale per ciascuno degli anni del prossimo triennio e 10 milioni di euro per il funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera. Infine voglio ricordare

nel campo della ricerca applicata in ambito navale. È un istituto che io invito i colleghi a visitare, perché è uno dei primi tre istituti in questo settore al mondo, che ha avuto riconoscimenti ricorrenti in ambito internazionale per la propria attività e che purtroppo viene a vivere una situazione di difficoltà che non merita e che va assolutamente superata. Ed ancora, si istituisce un fondo di 350 milioni di euro per l'anno 2007 e di 450 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 destinati a spese per il funzionamento dello strumento militare. Si dispone, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di 20 milioni di euro destinati al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione e manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate. Signor Presidente,colleghi, i 350 milioni di euro destinati all'esercizio non compensano certo i 1.400 milioni di euro di taglio effettuato con la finanziaria dell'anno scorso, viceversa, le risorse destinate agli investimenti sono superiori rispetto ai 1.076 milioni di euro di taglio effettuato lo scorso anno, raggiungendo quest'anno la cifra di 1.700 milioni di euro, e rappresentano una netta inversione di tendenza anche in considerazione della strutturalità dell'intervento che è previsto per l'esercizio nella misura di 450 milioni nel successivo biennio per ogni anno e di 1.700 milioni per quest'anno, di 1.550 milioni per il 2008 e di 1.200 milioni di euro per il 2009, per l'investimento. Come ha sostenuto il Ministro della difesa, sarebbero state necessarie, soprattutto nell'esercizio, per superare il *gap* creato negli ultimi anni, ulteriori risorse, ma siamo solo all'avvio di un oculato e indispensabile intervento per recuperare il taglio enorme di risorse realizzato nella scorsa legislatura a danno della difesa. Abbiamo oggi un aumento di 2.085 milioni di euro, che porta il bilancio relativo alla funzione difesa a circa 14.522 milioni di euro, rapporto tra risorse per funzione difesa e prodotto interno lordo che passa dallo 0,825 per cento a oltre lo 0,95 Il rapporto tra le spese per il personale e lo stanziamento per la funzione difesa, dopo queste correzioni, scende dal 72 per cento al 62 per cento, ripristinando rapporti dunque più adeguati tra le varie componenti del bilancio della difesa, cioè personale, investimenti ed esercizio, che, secondo il parere di tutti gli analisti, dovrebbe consistere nel dedicare il 50 per cento al personale ed il resto alle altre funzioni. I fatti dimostrano quindi che questa maggioranza, nonostante la situazione ereditata, è stata attenta alle problematiche di questo delicato settore ponendo attenzione sia al personale, sia a risollevare quei settori relativi all'esercizio ed agli investimenti penalizzati dal precedente Governo. Il risultato già è presente nell'inversione di tendenza e siamo certi che conseguiremo gradualmente un riequilibrio globale, in modo tale che gli impegni assunti per portare l'Italia, nel contesto internazionale, ad un ruolo adeguato al posto che occupa siano conseguiti, correggendo così quello che Berlusconi non ha concretamente fatto, pur avendo promesso che avrebbe portato le risorse per la difesa ad un livello in linea con i principali Paesi europei. È dunque paradossale che chi, fino alla fine della scorsa legislatura, dava giudizi positivi

di nasconderli, esprima oggi critiche alla linea di evidente e deciso recupero di risorse in questo fondamentale settore, considerato che la difesa e la sicurezza sono beni essenziali per qualsiasi futuro di progresso e sviluppo del nostro Paese. Voteremo, dunque, a favore invitando il Governo a risolvere anche nuove questioni insorte, quali quella del provvedimento, non ricompreso nel maxi emendamento, necessario per il personale civile della base USA *Navy* dell'isola di Santo Stefano nell'arcipelago della Maddalena.

Signor Presidente, nel gran vociare mediatico su questa o quella specifica misura contenuta nella legge finanziaria ha finito con offuscarsi, a mio giudizio, il profilo netto delle alternative in campo: la legge finanziaria del Governo di centro-sinistra, così come risulta dalla conferma delle sue architravi (come ama dire il Ministro dell'economia, che saluto e ringrazio per la sua presenza) e dalle profonde modifiche dei suoi interventi specifici, così come prodotti durante la lettura parlamentare;

creato dall'aumento delle entrate che si sta registrando, rispetto al 2005, nel 2006? Confesso, colleghi della opposizione, di non aver capito perché il centro-destra, al fine di rendere più chiara questa sua proposta alternativa, assolutamente legittima e proponibile, non abbia concentrato il fuoco della sua polemica sul bilancio di previsione a legislazione vigente.

la proposta di legge finanziaria; presenti una nuova Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico finanziaria, che registri l'aumento delle entrate che si sta realizzando nel 2006. nel 2006. Solo a quel punto, il Governo presenti una nuova Finanziaria, dentro i nuovi saldi definiti dalla nuova Nota di aggiornamento, e venga in Parlamento per discuterla. Che senso ha, colleghi dell'opposizione, sostenere questa linea e non partecipare poi alla discussione sul bilancio di previsione a legislazione vigente? Tralasciamo i misteri delle tattiche parlamentari e veniamo alla sostanza. Sono credibili le basi di questa linea alternativa del centro-destra?

Rispetto al 2005, le entrate stanno crescendo in modo significativo, tanto che - a legislazione fiscale del centro-destra perfettamente vigente,

al valore del 2001. Seconda considerazione. Si può concludere, già oggi, che le entrate 2006 saranno non solo superiori a quelle del 2005 - questo è assolutamente certo

Ma, ciò che conta è proprio rispondere correttamente a questa domanda. Siamo tutti d'accordo sul fatto che le entrate 2006 stanno superando quelle del 2005 in modo molto significativo, tant'è che la pressione fiscale

I numeri veri, che si desumono guardando le tabelle, e soprattutto guardando il bilancio assestato a legislazione vigente - suggerisco questo esercizio ai colleghi del centrodestra (non mi sembra troppo complicato) - consigliano una risposta più articolata. La mia risposta è la seguente. Forse, quando i dati di cassa oggi disponibili consentiranno trasposizioni sulle entrate di competenza e sarà fra qualche tempo -, le entrate 2006 si avvicineranno alle previsioni più di quanto in passato si siano mai avvicinate.

le entrate 2006 saranno superiori di gran lunga alle previsioni assestate 2006. Naturalmente, speriamo che lo siano. Mi accontenterei comunque che si avvicinassero, perché oggi i dati a nostra disposizione attestano di una notevole distanza. Escludo quindi che, già oggi, si possa concludere che queste entrate supereranno certamente le previsioni. colleghi dell'opposizione, si pone un problema rispetto alla vostra linea. Il bilancio di previsione, infatti, ha una nota caratteristica: le previsioni di entrata scritte nel bilancio coprono previsioni di spesa. Quindi, se guardiamo al bilancio 2006 e guardiamo all'andamento delle spese, dobbiamo cercare di indagare se questo aumento prevedibile delle entrate a consuntivo 2006 rispetto al 2005 sarà tale da colmare le previsioni al punto tale da chiudere la forbice rispetto alle previsioni di spesa 2006, che sono quelle assestate e che hanno un livello di certezza, purtroppo, decisamente più elevato.

la terza domanda è la seguente: quante delle maggiori entrate 2006 possono essere credibilmente trasferite nel bilancio di previsione 2007, a legislazione vigente - ecco perché vigente - ecco perché sono stupito della vostra scelta di non discutere il bilancio di previsione a legislazione vigente - cioè prima dell'intervento della legge finanziaria che, come è noto, modifica le tabelle del bilancio, modificando la legislazione vigente? Il centrodestra risponde con sicurezza che almeno 25 miliardi di queste entrate sono trasponibili nel bilancio a legislazione vigente per il 2007. per il 2007. A mio giudizio, se seguissimo la scelta implicita in questa risposta compiremmo una scelta pericolosa per la stabilità della finanza pubblica, pubblica, per il merito di credito di un Paese molto indebitato come il nostro e, quindi, per la stabilità dell'intero sistema economico italiano. Dico questo per due ragioni molto semplici. La prima: le entrate 2006 -onorevoli

e positività), fanno registrare un'elasticità alla crescita del prodotto interno lordo del tutto anomala rispetto alla serie degli anni precedenti.

A proposito, ho notato incredibili emendamenti che aumentano di qualche milione di euro il fondo ordinario per l'università

non ignorare l'aumento del gettito 2006 (ci mancherebbe altro!), ma proiettare nel 2007 l'aumento del gettito solo nei limiti dell'elasticità alla crescita del prodotto interno lordo di operare una correzione strutturale dei conti pubblici, interamente concentrata nel 2007 - lo sottolineo anche ai colleghi della sinistra antagonista della nostra coalizione

stilando un bilancio 2007 che, per la prima volta dopo molti anni, rispetta quelli che gli economisti chiamano la «regola aurea». Da anni il bilancio italiano non rispetta la regola che vuole che lo Stato, sì, possa indebitarsi, ma lo faccia per spese in conto capitale. Bene, do una notizia: il bilancio 2007, con questa finanziaria, rispetta la regola aurea, ciò che i bilanci Italiani (non solo quelli del centro-destra, ma anche una parte significativa di quelli del centro-sinistra) non fanno da molto tempo. Questa linea, a nostro avviso, corrisponde meglio agli interessi di questo

Se il problema è questo, l'infrastutturazione del sistema attraverso la spesa in conto capitale è un nodo strategico, che - malgrado il volume globale del debito - dobbiamo essere in grado di affrontare.

molte contraddizioni e, soprattutto, molte carenze ed assenze. Bene, signor Ministro, Lei ha ragione di rivendicare il fatto che le architravi siano rimaste quelle che erano; se mi permette una valutazione critica, però, a mio avviso, non ha ragione quando afferma che la legge finanziaria è ancora ancora quella: non lo è, perché è stata profondamente modificata, per chiudere quei vuoti e per intervenire con politiche specifiche che ne rafforzano l'ispirazione di fondo. Credo che questo sia un giudizio più fondato.

1 - non a caso, votata anche dall'opposizione, con la sola eccezione dell'UDC - la quale collega all'aumento del gettito prevedibile

che affrontano, uno dopo l'altro, tutti - e dico tutti! - i problemi posti dal variegato mondo della piccola impresa italiana (dagli studi di settore all'apprendistato, per arrivare fino alle norme per la successione d'impresa).

abbiamo fatto ciò che questo mondo ci chiedeva, laddove ci domandava cose giuste, che abbiamo condiviso. In terzo luogo, abbiamo realizzato interventi che mettono in bilancio le risorse necessarie per aprire la stagione contrattuale del personale di pubblica sicurezza. I fondi per la specificità contrattuale di tale categoria non c'erano (ma adesso vi sono, e questo apre la possibilità per il rinnovo contrattuale); così come

introdotto la compartecipazione dinamica all'IRPEF per gli enti locali: l'architrave del federalismo fiscale, attuativo dell'articolo 119 della Costituzione. Non c'era e adesso c'è. Infine, quinto punto, con un intervento di riforma strutturale della macchina pubblica abbiamo disposto l'unificazione delle scuole di alta formazione della pubblica amministrazione e abbiamo messo fine allo scandalo di Sviluppo Italia, con una norma che la ristruttura profondamente e in modo radicale.

Si è aperto nel centro-sinistra il dibattito sul dopo finanziaria: in un brutto linguaggio politichese si parla di «fase 2» oppure di correzione di rotta, di cambio di passo o di accelerazione, di integrale rispetto del programma (un'espressione un po' talmudica messa così), ovvero di Topolino, definizione adottata l'altro giorno da uno dei due vicepresidenti del Consiglio. Per non prendere partito e anche per cercare di usare un linguaggio comprensibile ai più, dirò che il tema vero riguarda ciò che la maggioranza e il Governo dovranno fare il prossimo anno, quindi parliamo di anno 2007 del Governo, del giorno dopo la finanziaria che stiamo per approvare. Il punto di partenza non può non essere il riconoscimento del momento molto difficile che il Governo sta affrontando nel rapporto con il Paese. Limitarsi a parlare di difetti di comunicazioni o a dire che il popolo prima o poi capirà sarebbe prova di arroganza. Nel momento in cui giunge a conclusione l'*iter* della legge finanziaria, bisogna anche dire che io non credo che i problemi della maggioranza siano nati con la legge finanziaria, risalgono a prima, e i limiti della finanziaria ne sono semmai una conseguenza, non una causa. Questo punto è importante perché altrimenti si rischia di commettere errori di analisi. Il risultato delle elezioni politiche è stato quello che è stato: non sarà ricorrendo a presunti brogli, che non esistono, e neppure illudendosi con conti e riconti dei voti, come si illude e illude l'ex Presidente del Consiglio, che il risultato potrà essere modificato. Il tema per noi è un altro, ed è che il centro-sinistra ha vinto con poche migliaia di voti. In democrazia questo conta ed è più che sufficiente per un Governo di legislatura, ma il tema che dobbiamo discutere nella maggioranza è la ragione di un risultato così inferiore alle aspettative. Solo errori di campagna elettorale, senatore Boccia, che pure ci sono stati, solo difetti di direzione politica in quella fase, che pure ci sono stati? è anche, io credo, una insufficiente comprensione dell'Italia così come è davvero, non come la si immagina a tavolino, dei suoi veri problemi, di quelli del mondo produttivo, così come di quelli dei ceti popolari, della classe operaia, degli intellettuali che operano nell'università, nella ricerca, nelle professioni. È da qui che occorre ripartire, così come occorre ripartire dalla richiesta degli italiani di ogni parte politica di un profondo e serio rinnovamento della politica. Il primo atto del nuovo Governo, la moltiplicazione degli incarichi di Ministro e di Sottosegretario, male è stato accolto dai cittadini e per di più, per la confusa sovrapposizione di competenze e di funzioni che ne è derivata, ha determinato conseguenze negative sull'azione di Governo di cui abbiamo visto anche nella legge finanziaria e anche qui in Senato gli effetti negativi. È venuto poi l'indulto: un giusto provvedimento di clemenza in via di principio, approvato del resto da gran parte del Parlamento. Ma i colleghi sanno perfettamente, per avere vissuto le ventiquattro ore durante le quali il Senato è stato costretto a luglio a votare quella legge, che il contenuto, sbagliato nel merito (non nel principio, lo ripeto) di quella legge è stato deciso fuori dal Parlamento, in vertici tra partiti di maggioranza e di opposizione.

Questo discorso riguarda anche l'opposizione, che deve decidere se continuare a condurre una sterile opposizione in attesa dell'improbabile spallata, oppure concorrere al lavoro parlamentare. Abbiamo dimostrato che lavorare insieme è possibile

dopo le significative prese di posizione dei *leaders* dei due maggiori partiti di opposizione, l'onorevole Fini prima, l'onorevole Berlusconi poi. Poi è arrivata la legge finanziaria, una legge di enormi dimensioni quantitative in termini sia di miliardi di euro, sia di migliaia di norme giuridiche. A quest'ultimo proposito, per quanto mi riguarda, su questo secondo aspetto sono molto vicino ad un caso di coscienza: dobbiamo essere tutti consapevoli - l'attuale opposizione per ciò che ha fatto nella passata legislatura, noi per il presente - che vi è un'alterazione non lieve dei princìpi costituzionali in materia di funzione legislativa delle Camere. parlato di coscienza e, come si sa, la coscienza per ciascuno - come è naturale che sia per gli esseri umani - ha profili diversi: per qualcuno sono decisivi i grammi di *cannabis*, per altri i princìpi della democrazia parlamentare. Mai più una finanziaria come questa, dal punto di vista istituzionale. Certo, il sistema va riformato - se ne è parlato benissimo in vari interventi, fra cui quello del senatore Morando - e lo si ripete periodicamente, ogni anno. Se si deve riformare si riformi, ma è del tutto chiaro che vi è anche un problema politico. Se una finanziaria esce dal Governo con oltre 200 articoli, se dal giorno successivo i Ministri protestano e propongono modifiche, se il Governo non tiene conto della volontà della maggioranza parlamentare - come è accaduto per più aspetti del maxiemendamento - il problema non è istituzionale. Eppure, attraverso il mirabile lavoro condotto in Senato dal Presidente della Commissione bilancio, dal relatore e da tutti i senatori, si era arrivati molto vicini alla possibilità per il Governo di tener conto della volontà effettiva della maggioranza parlamentare. In queste circostanze dare la colpa al sistema, che pure - ripeto - va cambiato, è quanto meno eccessivo. Da ragazzino ogni volta che succedeva qualcosa si dava la colpa al sistema; più tardi ho capito che forse, anche con il sistema così com'è, si può cercare di fare di meglio. Mi sarei permesso di dire al ministro Padoa-Schioppa, se ci avesse degnati di maggiore tempo a sua disposizione, e glielo dico attraverso i lavori parlamentari,

Sono, infatti, venute dal Governo misure delle quali al posto del ministro Padoa-Schioppa non mi sentirei di rivendicare orgogliosamente la paternità. Mi riferisco al tentativo - poi sventato - di introdurre un piccolo *spoils system ad personam* nel suo Ministero, alla scandalosa norma che ha eliminato ogni tetto retributivo per i *manager* d'oro e ha anche attribuito loro - unici lavoratori in Italia - la scala mobile sotto forma di aumento automatico della retribuzione ogni anno parametrata all'inflazione (resti a verbale che non è questo che la maggioranza aveva chiesto); mi riferisco alla norma sul tetto retributivo ai dirigenti pubblici manipolata nel testo che mi vedeva primo firmatario con un richiamo criptico, ma ben compreso da chi ha scritto la norma, cioè la restrizione di quel tetto solo ad un numero limitato di dirigenti. In compenso, vi è una grande e positiva riforma che riguarda i dirigenti di prima fascia in questa finanziaria: i più alti in grado potranno finalmente volare in prima classe e non stare con i comuni mortali. Ma è mai possibile che, nel momento in cui si chiedono sacrifici al Paese, vi sia una categoria che non solo dai sacrifici è esentata ma che addirittura si vede riconosciuti nuovi privilegi? Su questo tema voglio qui rivolgere un chiaro appello al presidente del Consiglio, Romano Prodi: la riduzione dei costi impropri della politica fa parte del programma dell'Unione, sul quale abbiamo chiesto i voti: lui e tutti noi. Ancora non ci siamo! Come si vede, non vi è solo la scandalosa norma sul colpo di spugna per le responsabilità davanti alla Corte dei conti. Apprezzo che il Gruppo di cui facci**o** parte abbia preso all'unanimità e con grande determinazione l'iniziativa di chiederne l'abolizione, prima che essa possa produrre i suoi effetti potenzialmente devastanti. Ma resta il problema di chi e perché ha deciso di introdurre quella norma. Non mi interessano le ricostruzioni dietrologiche. Il problema che pongo è un altro e su questo chiedo una risposta dal Governo: come è possibile che in un Governo come il nostro vi sia stato qualcuno che ha pensato di introdurre una norma che purtroppo ricorda quelle del Governo Berlusconi - del quale ha abbondato - contro le quali tanto e giustamente abbiamo protestato nella passata legislatura? Ripeto al Presidente del Consiglio: Romano, batti un colpo! La via maestra per recuperare un consenso dei cittadini è dimostrare che i politici, nel momento in cui chiedono sacrifici agli italiani, siano in grado di realizzare non dico sacrifici perché questa parola mi sembrerebbe offensiva rispetto alle sofferenze di tanta povera gente - ma almeno un autocontenimento, un limite alla nostra ingordigia e alla nostra arroganza. Al ministro Giuliano Amato, che recentemente si è accorto del rischio di populismo di destra, vorrei dire che in altri Paesi europei come l'Austria e l'Olanda il populismo è stato sconfitto da moderne forze di sinistra, socialiste e socialdemocratiche, con una seria azione riformatrice, attenta alle esigenze del mondo del lavoro e dei settori produttivi e, soprattutto, attenta ad ascoltare e a cercare di dare una risposta, le risposte proprie di una moderna sinistra riformista, alle domande che quelle spinte populiste e reazionarie esprimevano. Affrontiamo allora in questo anno 2007 i problemi del Paese, come sono avvertiti dalla gente comune: per la gente comune, il problema sono le pensioni da fame che purtroppo ancora oggi molti italiani hanno e le pensioni da fame che avranno i giovani chiusi nel buco nero del precariato e della disoccupazione. Non riproviamo a mettere i padri contro i figli. Ci è costato già nel 2001 una pesante sconfitta elettorale! Problemi veri del Paese significa porsi il tema del carovita, della povertà, per il quale non bastano manovre sulle aliquote. Oggi un operaio, un lavoratore che guadagna 1.000 euro al mese, se non ha altri redditi in famiglia è povero. La redistribuzione fiscale non basta più in un sistema come il nostro, dove vi è un meritorio impegno di questo Governo contro l'evasione fiscale. Ma il sistema ha le caratteristiche che ha. La tutela dei più deboli si fa con i servizi pubblici, con i diritti sociali, con ciò che è rimesso in discussione dai fautori dell'unica ideologia che è rimasta nel nuovo millennio: l'ideologia del neoliberismo, del monetarismo, del mercato come nuovo idolo. Tra i segnali positivi dei miglioramenti introdotti dal Senato, ai quali giustamente faceva riferimento il collega Morando, vorrei aggiungere e dare particolare rilievo all'avvio del piano di stabilizzazione dei lavoratori precari della pubblica amministrazione; una misura che, secondo un sondaggio pubblicato oggi, convince i tre quarti degli italiani - non credo siano tutti precari della pubblica amministrazione - con buona pace dei fautori delle ideologie di cui parlavo. Bisogna investire maggiori risorse nella scuola, nella ricerca, nell'università pubblica non solo perché, come giustamente si dice, la qualità di un sistema e la produttività si esprime lì, ma anche perché nella ricerca, nella scuola e nell'università pubblica si combattono le disuguaglianze, in un Paese in cui ancora il figlio di un operaio ha dieci possibilità in meno del figlio di un laureato di arrivare a sua volta al titolo di studio superiore. Lasciamo che i ricchi ridano un po'! Tanto non saremo certo noi a farli piangere.

Nella Nota di aggiornamento del 30 settembre scorso e nella contestuale Relazione previsionale e programmatica per il 2007 si chiarisce, si ribadisce, anzi, si accentua una strategia di abbattimento del debito pubblico e si parla dell'obiettivo di scendere, a fine legislatura, se non ho inteso male, non più al 99 ma al 97 per cento. Per carità, sarebbe bello. Ma premesso che il parametro del debito pubblico, a differenza di quello del *deficit,* non è vincolante ai sensi del Trattato di Maastricht, mi domando, e domando al sottosegretario Giaretta: che cosa vuol dire questo in concreto nella prossima finanziaria? Forse un'altra cura da cavallo per abbattere di altri due punti nel 2007 il differenziale del debito pubblico? Eppure, è necessario lo sviluppo dell'economia. Nella stessa Relazione previsionale e programmatica si dice che lo sviluppo dell'economia italiana subirà un lieve rallentamento per effetto della manovra. Non sono un esperto in questo campo e mai come in questo settore cerco di esercitare la virtù dell'umiltà. Ho letto un libro di teologia - a volte capita, nel tempo libero - in cui si dice che la virtù dell'umiltà è fondamento di tutte le altre; chiedo però di esercitare la virtù dell'umiltà anche a chi siede nei banchi del Governo. Autorevoli personalità suggeriscono vie diverse. C'è un documento firmato da 60 noti economisti che indicano un'altra strada: non l'abbattimento, ma la stabilizzazione del debito rispetto al PIL. C'è il professor Giuseppe Guarino, già ministro del tesoro nel Governo Ciampi, che sta indicando in saggi interventi sulla stampa vie diverse: chiedo di discuterne. Onorevoli colleghi, il voto di fiducia chiesto dal Governo su questa legge finanziaria non è solo un dovere nei confronti degli elettori che mi hanno votato per sostenere questo Governo, è anche un segno di fiducia in senso proprio. senso proprio. Sempre quel teologo di cui parlavo prima diceva che la più giusta traduzione della virtù teologale della *fides* non è «fede», ma «fiducia». Non fede irrazionale, cieca e astratta, ma fiducia per continuare a credere, a credere che la seconda esperienza di centro‑sinistra non ripeta gli errori della prima: siamo quasi tutti gli stessi di allora, perseverare sarebbe diabolico.

Signor Presidente, colleghi senatori, nel mese di luglio il decreto Bersani-Visco è stato accolto da una vasta opinione pubblica come un provvedimento finalizzato alla liberalizzazione di risorse e di opportunità per consumatori e cittadini e di modernizzazione del Paese, una modernizzazione della quale è parte integrante e principio costitutivo una dura e severa lotta all'evasione fiscale. Non a caso, le resistenze e le proteste delle categorie interessate, che pure ci sono state e sono risultate assai aspre, non solo non hanno incontrato alcuna solidarietà da parte dell'opinione pubblica nel suo insieme, ma hanno anzi suscitato la preoccupazione che potessero interrompere il percorso di innovazione avviato dal Governo. Andrete fino in fondo o vi fermerete e magari tornerete indietro dinanzi alle resistenze corporative? Questa è la domanda che ci siamo sentiti rivolgere nel mese di luglio. Una domanda dalla quale emerge che i cittadini italiani hanno dimostrato di apprezzare le scelte segnate da dinamismo e innovazione, nella direzione della liberazione di energie, capacità e opportunità e che si aspettano da noi un metodo di Governo all'insegna del primato dell'interesse generale. È come se il Paese avvertisse che è solo per questa via che l'Italia potrà rimettersi in moto: basta particolarismi, basta egoismi corporativi, basta frammentazione degli interessi, basta guerra di tutti contro tutti e basta, a maggior ragione, con una politica che si limiti a riflettere o addirittura finisca per amplificare la frammentazione corporativa della società, con la perenne conflittualità tra partiti della stessa coalizione, talora perfino tra Ministri dello stesso Governo. Per salvarsi della decadenza e dal declino, l'Italia ha bisogno di riforme incisive e profonde e non c'è riforma possibile senza la coesione, la solidarietà e l'unità vera tra le forze riformatrici. Se la politica non riesce ad esprimere la necessaria, disciplinata tensione verso l'obiettivo del cambiamento, nella società si diffondono la sfiducia, il disincanto e la rassegnazione. Non si coglie più il nesso tra la politica e l'interesse generale; aumentano le derive centrifughe e le spinte particolaristiche; governare in un contesto nel quale non si può solo galleggiare diventa allora impossibile. Se vogliamo guardare in faccia la realtà e chiamare le cose con il loro nome, questo è il pericolo che stanno correndo il nostro Governo e la nostra maggioranza in questi mesi: il pericolo di una crisi di fiducia nel rapporto con il Paese, del quale si sono visti segnali preoccupanti nel corso del lungo *iter* della finanziaria. È stato il presidente Ciampi il primo a suonare l'allarme: disse subito di stare attenti perché non si coglieva il senso di una missione per il Paese. Per usare un'immagine del senatore Morando, potremmo dire che non si coglie la foresta, si vedono solo gli alberi. Non si ci si può impegnare su una manovra straordinaria per portata quantitativa, una manovra che finisce per colpire innumerevoli grandi e piccoli interessi particolari, se il Paese non ne comprende il significato complessivo e generale. In effetti, la legge finanziaria presentata dal Governo, e poi profondamente trasformata dal lavoro parlamentare, in particolare qui al Senato, è tutt'altro che di ordinaria amministrazione ed è segnata, cari colleghi dell'opposizione, da una netta discontinuità rispetto alla linea della passata legislatura. Nella passata legislatura la politica economica di Berlusconi e Tremonti ha dato all'Italia la crescita zero mentre l'economia mondiale conosceva la fase di sviluppo più impetuoso nella storia recente, il dissesto dei conti, con tre punti di PIL di spesa corrente in più, l'azzeramento dell'avanzo primario, la ripresa del debito e un grave aumento delle disuguaglianze. Le vaste critiche a questa finanziaria, non tutte infondate come abbiamo riconosciuto (in particolare nel dibattito in Commissione, cari colleghi dell'opposizione), sarebbero state più credibili se vi foste chiesti dinanzi al Paese perché non siete riusciti in nessuna delle tre missioni che vi eravate proposti: il rilancio dello sviluppo che non c'è stato, il taglio della spesa che invece è aumentata e la riduzione delle tasse che, confrontando il livello della pressione fiscale del 2001 con quello del 2006, vediamo che neanche essa c'è stata. La finanziaria 2007 si propone allora di aprire un ciclo nuovo, orientato all'obiettivo di tenere insieme il risanamento finanziario con la ripresa dello sviluppo, in un quadro di equità sociale. Quelli che Prodi e il ministro Padoa-Schioppa hanno definito i muri maestri della manovra sono robusti e solidi (li ha già citati il presidente Morando): il disavanzo di bilancio, che oggi, con la sentenza sull'IVA e l'emersione del debito delle Ferrovie sfiora il 6 per cento, viene riportato in un anno sotto la soglia del 3 per la prima volta, il livello complessivo delle spese per investimento supera il livello dell'indebitamente netto dello Stato e ci sono misure significative sul terreno dell'equità. Questa finanziaria avvia, infatti, una redistribuzione di reddito a vantaggio prima di tutto di chi ha di meno, con una rimodulazione fiscale ispirata a equità sociale e con un impegno straordinario di riduzione dell'enorme massa di fisco eluso ed evaso. maxiemendamento, approvato dalla Commissione bilancio del Senato, che prevede di destinare la quota strutturale dell'incremento di gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale alla riduzione delle aliquote e a benefici in favore degli incapienti è la traduzione in impegno concreto dello *slogan*, gridato per decenni e mai realizzato, «pagare tutti per pagare meno».

in particolare con riferimento alla piccola impresa e al mondo del lavoro autonomo, che erano stati pesantemente penalizzati dalla prima versione della finanziaria e hanno trovato invece accoglienza alle loro richieste. Tuttavia, signor Presidente, ci troviamo di fronte ad una finanziaria che ha segnato una difficoltà nel nostro rapporto con il Paese; penso che questo tema non possa essere ignorato da una maggioranza e da un Governo che hanno davanti cinque anni di lavoro intenso e che non possono non prendere atto di questa difficoltà nei confronti del Paese. Credo che prendere atto di questa difficoltà nel rapporto con il Paese significhi, innanzitutto, proporre alla politica economica un vero e proprio rovesciamento di paradigma. L'Italia non è più in grado di reggere un conflitto distributivo tradizionale, da qualunque parte lo si voglia condurre. Questo è un punto che ancora, a livello politico, non siamo riusciti a capire da nessuna delle due parti, a me pare nemmeno dalla parte dell'opposizione, per la verità, ascoltando gli interventi in questo pur ampio dibattito. Dobbiamo prendere atto invece che l'Italia non è in grado di reggere un conflitto distributivo tradizionale, perché un Paese come il nostro, che da dieci anni cresce di un punto al di sotto della media europea, è un Paese nel quale tutti i settori della società e dello Stato sono in sofferenza e nessuno di essi può realisticamente pensare di alleviare la propria difficoltà aggravando quelle altrui. Sono in sofferenza tutti i settori pubblici, basta sentire il dibattito parlamentare nelle diverse Commissioni: dalla sanità alla giustizia, dalla sicurezza alla scuola, dalle infrastrutture alla ricerca, dagli enti locali all'assistenza, non c'è settore che non si percepisca come sotto finanziato e non domandi maggiori risorse. Tuttavia, senza un rilancio della crescita, è impensabile porre rimedio a questa condizione perché è impensabile sia una significativa redistribuzione orizzontale da un settore all'altro sia un ulteriore aggravio fiscale sul settore privato, dato che anche la pressione fiscale nel nostro Paese sta raggiungendo livelli critici. Del resto, se si confronta la percentuale di prodotto interno lordo che l'Italia destina ai vari settori di spesa pubblica e la si paragona con quella degli altri Paesi, si vede che la nostra quota è nella media europea, pur con l'anomala incidenza di una spesa per interessi sul debito che è quasi il doppio dell'area dell'euro. Sul versante privato la sofferenza non è meno avvertita e denunciata; non c'è categoria che non lamenti - per lo più non infondatamente - un eccesso di pressione fiscale che ne limita la competitività e che non chieda di privilegiare i tagli di spesa alle manovre sulle entrate. Ma abbiamo già visto che, in un contesto di crescita zero, se sono stretti i margini per l'aumento della pressione fiscale, non sono affatto più larghi quelli per una riduzione significativa della spesa. La verità è che l'inflazione da domanda di risorse pubbliche - vuoi nella forma di aumento della spesa, vuoi in quella di riduzione della pressione fiscale - copre il vero problema del Paese, che è il grave ritardo, accumulato negli anni, nella modernizzazione complessiva del nostro sistema economico e sociale. Un ritardo di modernizzazione che trova la sua espressione sintetica in quello che gli economisti chiamano l'indice di produttività totale dei fattori; da molti anni in costante calo relativo sulla scala mondiale. Un ritardo che è la principale ragione del vistoso rallentamento del nostro tasso di sviluppo. Il ritardo italiano ha radici molto profonde, lo ha detto il ministro Padoa-Schioppa nelle conclusioni che ha fatto nel dibattito in Commissione; è almeno dagli anni Settanta che il nostro Paese, esaurita la spinta competitiva che gli derivava dalla condizione di partenza, segnata da una pesante arretratezza economica e sociale, anziché imboccare con decisione la via della modernizzazione di sistema, ha preferito attardarsi a lungo nel limbo delle svalutazioni competitive del *deficit* pubblico. Una condizione pericolosa che ha alimentato inflazione e instabilità, fino allo *shock* del 1992; una condizione dalla quale il Paese è uscito solo con l'ingresso nell'euro. Attenzione, l'euro ci protegge dal rischio della crisi finanziaria e valutaria, ma non ci garantisce la crescita, anzi ci sottrae in modo definitivo i due principali strumenti che avevano alimentato la crescita drogata degli anni Ottanta: la svalutazione competitiva e il finanziamento pubblico in*deficit*. Per rimettere in moto la crescita c'è una sola strada segnata da due binari paralleli: il risanamento e le riforme. Dobbiamo procedere con determinazione sul binario del risanamento, perché dobbiamo liberarci dal cappio del debito che ci costringe ogni anno a bruciare una percentuale di reddito nazionale doppia di quelli degli altri Paesi europei per finanziare il debito pubblico, anziché anziché aumentare la spesa sociale, gli investimenti e ridurre la pressione fiscale. Ma con la stessa determinazione dobbiamo avanzare sull'altro binario, quello delle riforme, in due grandi direzioni: competitività del sistema produttivo, attraverso incisive misure di liberalizzazione dei mercati, e qualità, efficienza, produttività del sistema pubblico, a cominciare dai quattro macrocomparti di spesa: previdenza sanità, pubblico impiego, enti locali. Discuteremo col Governo l'apertura, che noi proponiamo e alla quale crediamo, immediatamente dopo l'approvazione della finanziaria, di una fase nuova segnata dal confronto sulle grandi dal confronto sulle grandi costellazioni che devono guidare nei prossimi mesi il nostro impegno di governo e politico-parlamentare: un tavolo per lo sviluppo, il lavoro, i redditi, la produttività, le liberalizzazioni e un tavolo per la modernizzazione e riqualificazione del settore pubblico. È in questo modo che potremo dare agli italiani la precisa sensazione che abbiamo raccolto il messaggio critico di queste settimane e lo abbiamo tradotto in un impegno rinnovato per il cambiamento del Paese. È in questa prospettiva, signor Presidente, che voterò la fiducia al Governo.

poco del proprio difeso e molto delle colpe degli altri significa che il proprio difeso qualche colpa ce l'ha. Le colpe di questa finanziaria sono tante e di più: è una finanziaria che si vuole proiettare in un aiuto al miglioramento della situazione economica e socioeconomica e che invece sta facendo aumentare, ben al di là,

che non ha, perché non ha certamente il merito dell'aumento del gettito fiscale. Si badi: mi riferisco al gettito fiscale, non a quella che in letteratura viene comunemente chiamata pressione fiscale. Perché quello che si è realizzato e a cui ha fatto riferimento il senatore Morando è un aumento del gettito per un allargamento della base contributiva.

dal senatore Morando e da altri a difesa della manovra finanziaria. Una manovra finanziaria che il senatore Morando, come tanti altri senatori della maggioranza, avrebbe dovuto studiare un po' di più, e d'altronde che non l'hanno studiata si vede, perché quando parlano di architravi, non ricordano che il ministro Padoa-Schioppa non parlava di architravi, parlava di mura maestre, quindi vogliono aggiungere qualcosa di più anche al lessico e alla capacità letteraria del ministro Padoa-Schioppa, non ricordando che non si può parlare di mura maestre e che queste mura sono soltanto del cartongesso e che al posto delle architravi vi è soltanto una soletta di casa rurale, perché tutto - siamo sicuri - franerà sull'onda della pressione popolare per una manovra che è assolutamente vessatoria. Che è vessatoria lo dicono anche gli stessi Ministri e gli stessi autorevoli senatori della maggioranza, nel momento in cui stamattina il senatore Viespoli parlava di «errori tattici»; gli errori, se sono tattici, si collocano fra gli errori della strategia, e ricordiamoci che gli errori della strategia, nella testuggine macedone, erano puniti dallo stratega stesso, che infilzava chi usciva dalla traccia della battaglia. Il vostro stratega sarà il popolo, perché il popolo vi punirà non già votandovi, ma non votandovi più, perché se economia politica significa organizzare risorse scarse, ripeto che di scarso in questo momento non ci sono le risorse, né l'organizzazione, ma di scarso c'è questo Governo.

ho ascoltato degli interventi precedenti che mi fanno pensare quale grande occasione mancata sia stata questa legge finanziaria, perché a mio parere a mio parere con essa è stata rappresentata in modo emblematico la crisi del nostro sistema politico e parlamentare. Abbiamo di fronte plasticamente una sorta di gigantismo del Governo, che ha esercitato una funzione esaustiva nel gestire questa materia così complessa e uno scomparire della funzione parlamentare, che è stata svuotata della sua ragione sua ragione essenziale: l'attività legislativa. La legge finanziaria, cioè il momento più rilevante della gestione, della programmazione, dell'azione di Governo, è stata concepita, gestita, mediata, formalizzata e perfezionata tutta nell'ambito del Governo e quando ascoltavo l'intervento brillante, anche se non sempre condivisibile, del presidente della Commissione bilancio, Morando, mi rammaricavo che quell'intervento fosse a commento commento della legge e non fosse il commento del protagonista di quella legge, perché quell'intervento doveva essere in qualche modo il punto di sintesi del processo parlamentare e della funzione che esso esercita. esercita. Se poi il risultato di questa alterazione del gioco istituzionale che, come ha spiegato bene il presidente Salvi, mette in discussione i postulati del nostro sistema costituzionale, eliminando dal campo dell'azione legislativa il Parlamento e riservando per intero al Governo tutto il processo, attraverso i meccanismi o dei decreti-legge, o delle fiducie, che sequestrano anche l'autonomia politica dei singoli parlamentari; se il risultato è quello di questa legge finanziaria illeggibile, indigeribile, inaccettabile, che mette insieme, accatastandoli interventi di rilevante portata che incidono su aspetti molto molto significativi dei rapporti economici e sociali interventi minuti, vorrei dire veramente di limitato contenuto, ma forse nei quali è possibile registrare il successo di qualche *lobby*, di qualche intervento magari a margine dei fogli che accompagnavano il documento finale; se il risultato è questo, siamo ben lontani da quanto auspicava, all'inizio della sessione di bilancio, il presidente della Commissione bilancio della Camera, l'onorevole Duilio. Egli diceva di augurarsi che la finanziaria 2007 fosse un documento stringato, essenziale nei suoi contenuti e nelle sue linee di fondo, coerente con gli obiettivi fissati nel DPEF di luglio, esteticamente presentabile, quanto a tecnica legislativa, dopo le brutture degli ultimi anni. Infatti: questo documento è perfettamente perfettamente aderente all'auspicio del presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati, onorevole Duilio. Ciò dimostra che l'imbarazzo è diffuso, che esiste una perfetta consapevolezza dell'impossibilità di fare ancora peggio,

tra Governo, Parlamento e anche la maggioranza parlamentare che sostiene il Governo. Gli imbarazzi, le critiche, le perplessità emerse nel corso di questo dibattito debbono interrogare il Governo, quantomeno alla pari con le incomprensioni caratterizzanti oggi il rapporto del Governo con la cittadinanza di questo Paese, con la distanza siderale - come è stato detto - tra questo Esecutivo e i cittadini italiani. italiani. La mia sensazione è che questo corto circuito, questa difficoltà così evidente non sia soltanto responsabilità di questo Esecutivo, inadeguato e presuntuoso, e nemmeno della condizione politica di questa maggioranza, che segnata da una conflittualità interna e da una lacerazione dei rapporti di alleanza che le impedisce di offrirsi al libero confronto parlamentare perché in questa sede vengano definite le soluzioni di sintesi (infatti, la Costituzione ha assegnato al ha assegnato al Parlamento il ruolo della sintesi degli interessi in campo con la definizione della norma come compromesso tra gli interessi; questo non è certamente accaduto). Certamente, su questa alterazione del gioco democratico incide l'interpretazione tutta italiana di un bipolarismo muscolare e forzoso, che impedisce un confronto libero e pacato, che sospetta chiunque assuma un'iniziativa in qualche modo irregolare perché lo schema costruito tende soltanto alla conflittualità permanente, ad un disconoscimento della legittimazione politica del proprio avversario.

Paese è privato di una linea di politica economica a lungo respiro, senza una politica delle infrastrutture strategiche condivisa e persino sulla politica estera

si è perduto in autorevolezza e competitività, entrando in una crisi strutturale del sistema economico e della nostra autorevolezza internazionale, situazione che interroga il futuro di questo Paese. Oggi, è necessario uscire da questo schema. Io avevo provato ad utilizzare in modo proprio la sede parlamentare offrendo un'iniziativa, anche rischiando il fraintendimento, rispetto a questo schema così rigido di appartenenze, per tentare di trovare una soluzione strutturale nuova al *deficit* di infrastrutture nel Mezzogiorno (di questo voglio parlare), immaginando una linea di finanziamento assolutamente originale per recuperare quella condizione di ritardo.

ma, se il deserto infrastrutturale è il Mezzogiorno, vi è la necessità di porre rimedio a questa condizione avendo un'idea forte. Avrei Avrei anche perdonato il Governo per questa iniziativa così invasiva sul terreno del prelievo fiscale, per questo intervento così forte, che interferisce anche sui processi di accumulazione legittima delle risorse dei singoli cittadini, se avesse avuto una *mission*, un orizzonte nel quale costruire una sfida per lo sviluppo e per la riunificazione nazionale. Qualche giorno fa la SVIMEZ ha celebrato i sessant'anni della sua azione consegnandoci un'ulteriore analisi

spaccato. Non si tratta più di divario, né di marginalità, ma di divaricazione. C'è un dualismo da combattere. Ci sono due Italie. L'Italia non è più soltanto lunga e stretta, come diceva De Gasperi, ma è anche spaccata nel livello delle infrastrutture, dei servizi e reddituale. Ci sono due Paesi che si stanno allontanando e le dinamiche segnano un'ulteriore divaricazione. Dov'é la sfida di questo Governo? L'avrei compreso se le risorse che sta accumulando sul terreno fiscale fossero impegnate in una grande battaglia che, per esempio, prendesse le mosse dall'analisi economica di un'associazione indipendente come la SVIMEZ.

straordinario perché si pensava che, se vi era una differenza così grande nel Paese, non poteva essere compito delle amministrazioni ordinarie porre rimedio a quella condizione. Si è costruito quindi l'intervento straordinario, abbandonato agli inizi degli anni '90 per le interpretazioni politiche, culturali, e che io mi permetto di definire antimeridionali: e non ho paura di tornare ad utilizzare questo termine, quando oggi in modo capzioso si prova a contrapporre una questione settentrionale a quella meridionale. Qui c'è una questione nazionale. Occorre accompagnare lo sviluppo, la competitività, l'innovazione delle aree forti del Nord del Paese, ma non si comprende che, se non si affronta in modo strutturale il tema del Mezzogiorno, questo Paese è destinato alla sconfitta. Infatti, nel Mezzogiorno c'è lo spazio vero per lo sviluppo, ci sono le risorse scolarizzate, ci sono gli spazi per le infrastrutture, c'è un mercato potenziale. Ci sono spazi di crescita quasi comparabili a quelli delle aree del Sud-Est asiatico, se si compie la scelta strategica di questo Paese che guarda, per esempio, alla cooperazione euromediterranea e alle prospettive di quel grande mercato potenziale, attrezzando questo territorio e scommettendo su di esso. princìpi di equità rigorosi, come quello di investire secondo il peso naturale, che è un parametro che tiene insieme popolazione e territorio. che vorrebbe dire che in questo Paese la spesa pubblica in conto capitale, quella che consente il governo del sistema, secondo le analisi macroeconomiche e senza evocare la cultura dell'intervento pubblico in economia, dovrebbe indirizzare il 60 per cento delle sue risorse al Centro-Nord e il 40 al Sud. Sapete a quanto ammonta l'investimento nel Sud? Al 26 per cento! Non soltanto, caro Governo, non colmiamo il divario, ma arretriamo ulteriormente nella nostra marginalità.

Se dovessimo misurare il quadro di risorse impegnate in tanti anni nell'assistenza generosa a un sistema imprenditoriale debolissimo del nostro Paese, fatto di finti capitali di impresa (che, però, possiede, ad esempio, i *mass media* e condiziona pesantemente il sistema delle comunicazioni), dovremmo interrogarci sui veri processi strutturali dell'economia; dovremmo capire quanto realmente interessa invertire alcuni processi, quanto sia equa

Nella finanziaria in esame, caro Presidente, in cui c'è di tutto, anche norme che non sono compatibili e che avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili dalla Presidenza, ci sono interventi incisivi e vorrei dire lesivi delle autonomie statutarie sul terreno della normazione di queste stesse realtà. in tre Regioni a Statuto speciale ci sono state modalità diverse di relazione del Governo centrale. Con la Regione Sardegna è stato ridefinito, riformulato tutto il sistema dei rapporti finanziari Stato-Regione, spero in modo vantaggioso per la realtà sarda; questa mattina, però, ho ascoltato il collega Massidda che era profondamente perplesso, non soltanto sul metodo seguito, ma anche sui contenuti di quel nuovo sistema di relazioni. Certamente la vicinanza politica e personale del *Premier* con il Presidente della Regione Sardegna ha consentito un'interlocuzione precedente, la definizione di un'intesa formale e il rispetto delle prerogative statutarie sarde. Qualcosa di simile è stato fatto anche con il Friuli-Venezia Giulia. Alla Regione Sicilia, che forse non è simpatica e certamente non è omogenea politicamente, è stato riservato ben altro trattamento:

di relazioni cordiali, un'intesa precedente. Non parlo dell'attivazione formale di un tavolo di negoziazione. Si norma, si interferisce, si incide e poi, con la forza di persuasione della potestà normativa già emanata, si pretende che la Regione sieda al tavolo della trattativa ed entro quattro mesi mesi accetti una ridefinizione delle norme di attuazione dello Statuto in materia di sanità, che ha un'incidenza enorme sulla spesa, con la spada di Damocle che, comunque, se l'intesa non viene trovata, l'effetto di aggravamento della quota di compartecipazione regionale sulla spesa sanitaria, che é comunque definita dal Parlamento nazionale con la legge finanziaria. È un aspetto non dico minimo, ma importante, che rivela anche il vizio di fondo di questa interpretazione dei rapporti Stato-Regione con la scarsissima fede che vi è nel sistema delle autonomie. Questo Governo non soltanto non ha cura della sostanza dei rapporti con i territori, in particolare con quelli più svantaggiati, ma neanche rispetta le forme costituzionali. Avrei voluto trovare, quella grande manovra di equità e riunificazione nazionale: allora, sì, avrei dato volentieri il mio voto a questo Governo, perché non mi sento vincolato da alcuno schema rigido di appartenenza. Ma

il mio voto contrario, nella speranza che il futuro possa rimodulare i rapporti e consentire di affrontare davvero una grande sfida di riunificazione nazionale.

Pensiamo, per esempio, a quanto è stato fatto, per la prima volta, per i precari: riteniamo che quello fosse un segno concreto perché restituiva tutela

a quella legge che ha massacrato il mondo del lavoro, la legge n. 30 del 2003, di cui vanno così fieri e orgogliosi i colleghi senatori del centro-destra, che non solo ha stravolto il mondo del lavoro, ma che ha

Abbiamo fornito anche un grosso contributo alla questione della scuola: 150.000 precari saranno assunti e resteranno aperte le graduatorie. Anche questo è un passo importante; non è esaustivo per il mondo della scuola, ma è un piccolo seme.

fa dire oggi che abbiamo riportato dei risultati. Mai come in questa fase, peraltro, il mondo agricolo non è soddisfatto: badate bene, non abbiamo risolto tutti i problemi, c'è ancora molto da fare, in particolare sul tema della ricerca scientifica

Certamente tutto questo non ci parlava di un profilo alto del Governo, aspettavamo ancora questo passo,

che ci sia ancora la possibilità del cambiamento, ma chiediamo al Governo che questo cambiamento ci sia realmente, che le persone possano dire che la loro vita sta cambiando, la loro, non quella che non vogliamo nemmeno guardare, perché l'abbiamo vista attraverso i vari panfili e tutto il resto.

le occasioni per affrontare questioni per qualcuno molto marginali, ma per me ed altri colleghi molto significative. Per quanto concerne la questione della portualità, l'autonomia finanziaria, così come è stata prospettata, è una falsa autonomia poiché non vi è capacità riconosciuta di contrarre mutui, ovvero emettere obbligazioni, per esempio, da parte degli enti territoriali. In secondo luogo, la nautica da diporto e la portualità turistica che in forza del decreto Burlando negli ultimi dieci anni ha compiuto passi da gigante riuscendo ad arrivare ad una equiparazione con la realtà europea grazie all'apertura - tra le tante cose - di 50 nuovi porti per la diportistica, e correlatamente cantieri per la costruzione di navi e barche, viene azzerata dal fatto che

quando con ogni probabilità, se questo stesso tipo di strategia fosse stata applicata anche agli *hub* di Genova e Trieste, per esempio, avrebbe assunto un significato ben diverso da quella incentrata, per l'appunto, sulla realtà di Gioia Tauro che, tra l'altro, ha dei bilanci in grave *deficit.* Ancora una osservazione a tale proposito. Si è parlato di riconoscere uno *status* di porto franco alla succitata realtà di Gioia Tauro *et similia*, ignorando come da oltre cinquant'anni vi sia uno *status* unico nel suo genere in Europa: il porto franco internazionale facente capo alla realtà dell'autorità portuale di Trieste che mai ha trovato piena attuazione. Concludo

grazie.